con cui si è espresso favorevolmente in merito alla realizzazione dell'insediamento militare americano nell'area dell'aeroporto "Dal Molin", ipotizzato nella zona posta ad est della pista aeroportuale. Tale parere è stato subordinato all'osservanza di talune condizioni, tra le quali l'assenza di impatti negativi sull'esistente aeroporto ed il mantenimento del suo attuale potenziale. A seguito delle molteplici perplessità espresse da vari esponenti politici e dagli imprenditori locali sull'impatto che la nuova struttura avrebbe potuto avere sull'ambiente circostante, soprattutto sotto l'aspetto della viabilità, e grazie all'azione di stimolo e proposta svolta dal commissario governativo Repubblica del 13 luglio 2007), è stata ritenuta più confacente all'interesse generale la soluzione progettuale che prevede la localizzazione dell'insediamento statunitense nell'area situata ad ovest della pista aeroportuale. Essa, infatti, recepisce le necessità manifestate dalle comunità locali ed elimina la gran parte delle ragioni di dissenso, anche di natura ambientale, che avevano accompagnato la scelta di ospitare l'esercito americano nel sedime aeroportuale vicentino. Le misure di mitigazione previste attenuano l'impatto dell'intervento e permettono la conservazione di aree di verde pubblico e di impianti sportivi, nonché l'utilizzazione di edifici già esistenti, consentendo anche di evitare modifiche alla viabilità cittadina. Il completamento a nord della circonvallazione di Vicenza rappresenta una delle misure di compensazione per remunerare i disagi eventualmente subiti dalla città. Tale soluzione progettuale alternativa, elaborata dai progettisti statunitensi, ha ricevuto il parere favorevole, all'unanimità, del COMIPAR (Comitato misto paritetico regionale) del Veneto, ai sensi della legge 24 dicembre 1976, n. 898, nella seduta del 19 novembre 2007, alla quale è intervenuto il sindaco di Vicenza, che ha espressamente manifestato la sua preferenza per questa soluzione, rispetto alla precedente localizzazione dell'insediamento. Anche le autorità statunitensi, sia a livello politico che a livello strettamente militare, hanno espresso il loro apprezzamento. La realizzazione dell'infrastruttura ad ovest della pista, pur se renderà necessaria la liberazione dell'area dalle attività italiane ora presenti, non comporterà affatto la demolizione di tutti gli edifici esistenti, ma solo di quelli - di un limitatissimo numero - ritenuti privi di valore architettonico, mentre saranno conservati, di intesa con la soprintendenza competente, gli altri. Il Ministero della difesa ha peraltro evidenziato la fattibilità tecnica del trasferimento delle funzioni svolte dall'Aeronautica militare entro il 30 giugno 2008. Inoltre, non è affatto prevista la definitiva demolizione della pista aeroportuale esistente, ma solo la sua rotazione e traslazione. L'ENAC, nel valutare tecnicamente fattibile la soluzione, con nota del 22 ottobre 2007, ha ritenuto che essa non pregiudica in modo sensibile le attuali, già purtroppo limitate, potenzialità di traffico dell'aeroporto. La limitatezza delle prospettive di sviluppo dello stesso, che - com'è noto - da tempo opera in costante e consistente perdita, ha indotto nella città di Vicenza un esteso dibattito sul futuro dell'infrastruttura, che non esclude la valutazione di migliori soluzioni infrastrutturali nel contesto territoriale limitrofo. Per quanto riguarda lo spostamento con rotazione e traslazione dell'attuale pista aeroportuale, si fa presente che, al di là delle problematiche operative, comunque temporanee ed inevitabili, connesse all'interferenza delle attività di cantiere, non si riscontrano palesi impatti negativi di natura permanente sull'aeroporto. Il predetto spostamento della pista, oltre a non presentare preclusioni di ordine tecnico - come evidenziato dall'ente competente - non pregiudica le prospettive di future attività dell'aeroporto più di quanto esse non lo siano attualmente per la sua configurazione attuale, in quanto «condizionato dalla sua collocazione in un contesto orografico complesso e dal carattere estremamente urbanizzato del territorio limitrofo». Anzi, si può addirittura sostenere che le modifiche alla viabilità e i miglioramenti progettuali potrebbero, al contrario, accrescere, seppur nei limiti di cui sopra, le possibilità di sviluppo dell'infrastruttura. La stima dei costi relativi allo spostamento della pista, comprensivi della parte di rifacimento, nonché di quelli delle eventuali demolizioni è attualmente in corso, dal momento che il commissario ha richiesto la previsione, bando, della mera evidenziazione dei costi stessi da parte dei concorrenti, onde possano essere scorporati e resi neutri rispetto al prezzo complessivo dei lavori di edificazione. In relazione all'addebito degli eventuali oneri subiti dall'aeroporto per l'inevitabile disagio in termini di interruzione e/o di rallentamento, dato dalla contemporaneità dei lavori (seppure dal punto di vista economico sia concretamente dubbio poter ravvisare oneri nella interruzione di un'attività che di per sé produce passivo), sono in corso i necessari accertamenti giuridici ed approfondimenti per verificare se ed a chi essi debbano fare materialmente carico. infine, presente che l'assemblea del consiglio di amministrazione della Società aeroporti vicentini ha rinviato le decisioni inerenti i costi dell'operazione ad una prossima riunione da convocare entro la fine del corrente mese.

ad alcuni in maniera soddisfacente, ma ad altri in maniera meno soddisfacente. Innanzitutto, devo dirle che dal punto di vista ambientale non mi pare che la scelta tra la parte occidentale e la parte orientale possa avere alcuna validità, perché il discorso ambientale era riferito ad un'utilizzazione da parte di una entità militare americana che rimane uguale da una parte e dall'altra;

tutta l'impiantistica di controllo e guida del volo, evidentemente se la parte americana si piazza ad occidente anziché ad oriente, che era completamente libero, dovrà essere prevista sia la ripulitura completa di quella parte, sia la smobilitazione di tutte le strutture che oggi consentono il volo. Il fatto che lo spostamento della pista possa non determinare una riduzione delle capacità di sviluppo operativo mi lascia invece assolutamente perplesso: questo non è vero, e voglio ricordare che parlo a nome di una città che è uno dei centri industriali, di rapporti internazionali e di esportazioni di primissimo piano, per cui certamente lo spostamento della pista non consentirà quegli sviluppi che la città

invece che lei avrebbe potuto comunicarli, fermo restando che essi sono in via di definizione, dato che la previsione di attribuzione del sostegno dei costi non richiede nessuna grossa analisi:

per eliminare tutto quello che ancora esiste nella parte dove si vuole far andare gli americani; sappiamo che ad un certo punto i lavoratori (naturalmente parlo anche a nome di quelli dell'aeroporto di Vicenza)

ricordare l*'iter* finora svolto circa la possibile individuazione dell'odontotecnico come professione sanitaria. L'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha prodotto profondi cambiamenti nel settore delle professioni sanitarie, in un'ottica dì armonizzazione con la normativa europea. L'obiettivo del legislatore è stato quello di disciplinare compiutamente le singole professioni e di accrescere il livello della formazione professionale, prevedendo sia corsi universitari, secondo una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale e secondo un modello formativo che comprende l'insegnamento teorico e un "apprendistato" pratico da svolgersi presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, sia ulteriori livelli di specializzazione (lauree specialistiche, *master* di primo e secondo Il Ministero della salute aveva individuato con propri decreti ventidue professioni sanitarie, per le quali, di concerto con i competenti soggetti istituzionali, venivano attivati i relativi corsi di laurea; in tale ambito, era stato inoltre previsto di ricomprendere tra le professioni sanitarie anche l'ottico e l'odontotecnico, già arti ausiliarie delle professioni sanitarie, predisponendo nel 2001 gli schemi di regolamento mirati a disciplinare le suddette nuove figure. Nel corso della attività istruttoria è stata più volte interpellata al riguardo la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCEO), la quale, relativamente allo schema di regolamento dell'odontotecnico, ha formulato alcune osservazioni, recepite in buona parte nel testo successivamente trasmesso al Consiglio di Stato per l'acquisizione del necessario parere. L'*iter* procedurale avviato è stato interrotto non per questioni di merito, concernenti le mansioni e il ruolo che l'odontotecnico avrebbe dovuto svolgere, ma a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che - com'è noto - ha modificato il riparto delle competenze normative fra Stato e Regioni. Per tali sopravvenute modifiche, infatti, l'individuazione di nuove professioni sanitarie non può più essere effettuata da parte dello Stato con atto avente natura regolamentare (come il decreto ministeriale), ma necessita di una norma di grado primario che, avendo individuato i princìpi fondamentali della materia, consenta alle Regioni l'emanazione della disciplina precettiva e di dettaglio. Conseguentemente il Ministero ha dato avvio alla predisposizione di una normativa mirata a disciplinare il settore conformemente alle nuove norme costituzionali. L'entrata in vigore della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che fissa i princìpi fondamentali in materia di professioni sanitarie e, in particolare, l'articolo 5 che disciplina la procedura per l'individuazione e la normazione di nuove professioni in ambito sanitario, ha indubbiamente posto fine ad una situazione di incertezza normativa. Desidero ribadire che la determinazione di avviare il procedimento per l'individuazione della professione sanitaria di odontotecnico costituisce una scelta di questa amministrazione, che ha tenuto conto delle caratteristiche specifiche di una professione la cui attività operativa si inserisce certamente nel contesto salute. Sottolineo che non è esatto quanto affermato negli atti parlamentari circa una possibile individuazione della professione sanitaria di odontotecnico con decreto ministeriale; infatti, nel rispetto dell'articolo 5 della legge n. 43 del 2006, tale individuazione avverrà al termine del previsto *iter*, mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepito in un decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri. Questa amministrazione, con nota del 9 novembre 2006, ha chiesto alla Conferenza Stato-Regioni l'indicazione dei rappresentanti regionali per la costituzione della commissione tecnica operante nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, come disposto dall'articolo 5, comma 3, della legge n. In data 11 luglio 2007 detta commissione ha espresso parere favorevole, suggerendo talune modifiche allo schema proposto, che sono state recepite dal Ministero della salute. Al fine di sottoporre alle valutazioni delle amministrazioni centrali lo schema di profilo professionale, si è svolta il 16 ottobre 2007 una Conferenza di servizi, nel corso della quale sono state accolte le osservazioni delle amministrazioni intervenute; in particolare, si è convenuto di prevedere specificatamente che l'individuazione della nuova figura professionale debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In data 13 novembre 2007 è stato richiesto l'assenso delle stesse amministrazioni all'ulteriore corso del provvedimento; successivamente a tale acquisizione si provvederà a sottoporre lo schema di accordo alle valutazioni della Conferenza Stato-Regioni. E' opportuno sottolineare che le attività attualmente svolte dall'odontotecnico, pur afferenti all'area della tutela della salute, non corrispondono a quelle svolte da altre professioni sanitarie; gli stessi operano nel campo delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie con metodiche operative che li pongono in stretto contatto con gli odontoiatri, senza, tuttavia, indebite invasioni di campo che, peraltro, laddove si verificassero, sarebbero comunque perseguibili per legge, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'odontotecnico. Pertanto, poiché le suddette metodiche non vengono modificate dall'*iter* normativo avviato, non è ipotizzabile alcuna parcellizzazione o invasione di competenze proprie di altre figure sanitarie. In merito al rilievo formulato negli atti parlamentari secondo il quale l'individuazione in esame sarebbe in contrasto con l'articolo 5 della legge n. 43 del 2006, il quale prescrive che le nuove professioni sanitarie debbano essere individuate in considerazione di fabbisogni connessi agli obiettivi di salute, previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute, il coinvolgimento della già citata commissione garantisce di evitare eventuali frazionamenti e sovrapposizioni con le professioni sanitarie già esistenti. Inoltre, va ricordato che fin dal 2001 il Consiglio superiore di sanità si era espresso positivamente sullo schema di decreto ministeriale, ravvisandone la rispondenza ad un effettivo fabbisogno del Sistema sanitario nazionale. In merito alle perplessità espresse circa la possibilità che, dopo l'individuazione delle nuove figure sanitarie, i soggetti in possesso dei vecchi titoli professionali verrebbero equiparati *ex lege* ai laureati, si segnala che per la nuova figura viene stabilito che i suddetti soggetti potranno svolgere l'attività professionale secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore delle norme relative al nuovo profilo. Del resto, secondo quanto previsto dalla normativa del 2006, l'equipollenza paventata non potrebbe realizzarsi se non con legge, mentre l'*iter* normativo avviato si concluderà con un decreto del Presidente della Repubblica. Va precisato anche che la formazione universitaria che gli odontotecnici dovranno avere corrisponde non ad una scelta discrezionale del Ministero della salute, ma alle disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992; in ogni caso la formazione universitaria non può, di per sé, essere considerata come fonte di indebite interferenze funzionali fra l'odontoiatra e l'odontotecnico, in considerazione della diversità, fra le due figure professionali, degli insegnamenti svolti, delle mansioni e del tipo di formazione. Non va sottovalutato, peraltro, che una formazione di livello universitario garantisce maggiori conoscenze professionali, a vantaggio della sicurezza dei cittadini e che, inoltre, una disciplina che definisce con precisione le caratteristiche e i contesti operativi degli operatori, risponde, fra l'altro, alla necessità di reprimere efficacemente il fenomeno dell'abusivismo; appare, pertanto, ragionevole sostenere che la regolamentazione della figura dell'odontotecnico risponderà positivamente a tali scopi. Da ultimo, si precisa che la direttiva comunitaria 93/42, citata negli atti parlamentari, si riferisce non alle professioni dell'area sanitaria, ma ai dispositivi medici, stabilendo le caratteristiche e i requisiti necessari per l'immissione in commercio. Va evidenziato che poiché gli odontotecnici già adesso realizzano e immettono in commercio dispositivi medici conformi alla normativa comunitaria, analogamente a quanto avviene per il tecnico ortopedico, il quale è un professionista sanitario,

Mi dichiaro soltanto parzialmente soddisfatto rispetto alle sottolineature che il Sottosegretario ha offerto alla nostra attenzione e cercherò rapidamente di spiegarne il perché. Nell'ambito della sua relazione, Sottosegretario, lei ha fatto riferimento a quelli che sono i princìpi legati alla normativa europea. Mi permetto soltanto di rilevare alla sua attenzione come all'interno dell'Unione Europea

di questo profilo ci porterebbe come Paese ancora, per l'ennesima volta, al di fuori della normativa comunitaria, con un evidente rischio di una procedura d'infrazione, che a questo punto sarebbe particolarmente evidente. Su questo piano, tra le altre cose, lei ha fatto un esempio collegato al mondo dell'ortopedia; lei sa meglio di me che in questa chiave il mondo degli odontotecnici da anni va sviluppando, a differenza degli operatori ortopedici, non solo una politica di affiancamento, ma in alcuni casi addirittura di sostituzione attraverso l'abusivismo dell'odontoiatra stesso. Gli esempi, sotto questo aspetto, sono illuminanti; tendono naturalmente ad interessare in maniera indiretta gli Ordini dei medici ed in maniera diretta poi le procure della Repubblica, sul piano più complessivo rispetto alle tante denunce che sono state formulate in questi anni. anche perché, al di là di 50.000 professionisti odontoiatri all'interno del nostro Paese, esiste un numero significativo di circa 23.000 odontotecnici, inseriti in circa 5.000 laboratori che operano - usiamo questo termine - a fianco, non sempre perfettamente in linea, rispetto al lavoro dell'odontoiatra stesso. Sul piano del percorso istituzionale,

in quanto la definizione delle nuove professioni di natura sanitaria necessita di funzioni che devono essere sviluppate - lo ha sottolineato anche lei nel suo intervento - evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con professioni già riconosciute e con le specializzazioni stesse.

(agli ambientalisti, ai chimici, ai biologi), mentre invece la centralità della professione medica resta, a nostro avviso, il vero punto di riferimento. Naturalmente, onorevole Sottosegretario, seguiremo con la debita attenzione debita attenzione gli sviluppi di questa situazione, convinti come siamo che l'allineamento della professione di odontotecnico a quella di odontoiatra resti un pericolo che deve essere evitato nel nostro Paese.

le informazioni che potrò fornire sono quelle pervenute dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che ha certificato che effettivamente il personale della Polizia penitenziaria in ha dovuto far fronte ad un periodo di gravoso lavoro per il concomitante verificarsi di una serie di circostanze ed esigenze operative. Infatti, nel mese di maggio 2007 è stato necessario impiegare numerose unità del medesimo personale sia in attività addestrative, sia in esercitazioni di tiro a fuoco. Contemporaneamente sono state presentate ben sei richieste di aspettativa speciale per la candidatura alle elezioni amministrative, mentre sono risultati assenti, a vario titolo, 33 unità di personale di Polizia penitenziaria. Allo stato, inoltre, tre unità risultano essere in servizio di missione, tre sono a disposizione del Centro militare ospedaliero, tre sono state distaccate per mandato amministrativo e altre 14 sono attualmente distaccate a vario titolo. Alla luce di tali chiarimenti, è evidente che l'impiego della Polizia penitenziaria in turni di otto ore, così come la mancata fruizione dei riposi anche programmati, è stata motivata dall'ineludibile esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza nell'istituto di Biella. Del pari si deve considerare la decisione di stabilire presso l'istituto di Biella un orario di turnazione di otto ore per alcuni posti di servizio deve essere garantita anche nel rispetto della tutela dei diritti soggettivi del personale di Polizia penitenziaria. In ogni caso, tutte le prestazioni di lavoro straordinarie sono state sempre eseguite previa acquisizione del consenso del singolo dipendente. Attualmente la situazione degli organici degli istituti penitenziari è seguita dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nell'ambito di questa attenzione si inserisce, per ultimo, il provvedimento di assegnazione di 450 agenti di Polizia penitenziaria destinati esclusivamente alle sedi settentrionali. Alla Regione Piemonte è stata destinata un'aliquota di 82 unità di personale di Polizia penitenziaria; il provveditorato regionale, nel ripartirla in modo da fronteggiare le esigenze più urgenti, ha destinato otto unità alla Casa circondariale di Biella. Quanto, infine, alla questione riguardante l'attività trattamentale effettuata nella sezione ad elevato indice di vigilanza dell'istituto di Biella, appare doveroso sottolineare che la stessa, così come è riferito dal provveditore regionale del Piemonte, si è concretizzata in un corso su *personal computer* della durata di un mese, al quale hanno partecipato complessivamente 10 detenuti. Il provveditore ha comunque messo in risalto che la realizzazione dell'iniziativa trattamentale è stata promossa da un'agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte, la Isvor FIAT, e che la sorveglianza delle attività formative non ha in alcun modo compromesso i diritti soggettivi del personale, essendosi utilizzate quattro unità di personale rese disponibili a seguito della simultanea chiusura per ristrutturazione di altra sezione detentiva

La risposta agli atti di sindacato ispettivo da parte del signor sottosegretario, avvocato Li Gotti, viene fornita lo stesso giorno in cui il Presidente del Consiglio assume l'*interim* del Dicastero della giustizia dopo le dimissioni del ministro Mastella

e che riguardano, così come lei ha avuto occasione e modo di vedere in Senato, i disagi e le difficoltà del Corpo degli agenti di custodia che vivono ormai una vita da reclusi tra i reclusi, impegnati nell'assolvimento di un servizio pubblico nelle difficoltà quotidiane, che vanno dalle piccole alle grandi cose. Mi sarei quindi aspettato, ad esempio, qualche elemento di valutazione rispetto alla questione posta posta anche relativa allo stato di disagio esistente nelle carceri e nel personale e ai numerosi suicidi che si sono registrati sulla fine del mese di dicembre, ben quattro, di cui due nel carcere di Marassi. quindi, di dare ogni ausilio a questo personale, anche psicologico, per una professione difficile, svolta in un ambiente particolare, privilegiando l'aspetto umano e il rispetto della persona.

al Piemonte; proprio in Piemonte si è registrata una qualche difficoltà operativa, perché molti penitenziari erano sotto organico e venivano a mancare gli elementi essenziali per poter svolgere questi compiti, soprattutto con gestioni discrezionali anche da parte del Consiglio regionale di disciplina, che si ripercuotevano negativamente sul Corpo. Abbiamo posto e riproposto numerose interrogazioni, e credo che qualche risultato l'abbiamo determinato.

Questo conferma la gravità di una situazione che richiede attenzione. Come dimenticare, poi, onorevole Sottosegretario, i tagli operati nella finanziaria, la mancanza di risorse economiche, la mancanza di remunerazione dello straordinario dovuto al personale, nonostante questo sia stato richiesto per assicurare compiti istituzionali. È una situazione, Presidente,

che su tali questioni, senza *vis* polemica, ci sia un atteggiamento da parte dell'amministrazione penitenziaria in grado di tener conto anche di questo personale che vive e soffre una situazione così difficile. La

Signor Presidente, la vicenda posta dalla senatrice Rame è estremamente complessa. Il tribunale per i minorenni di Firenze, il 9 settembre 2005, dopo aver rilevato che il minore G. S. mostrava forti segni di disagio, revocava l'affidamento del minore al padre S. T., incaricando il responsabile del servizio sociale competente di collocarlo presso una famiglia idonea. indicava, quale famiglia idonea, quella che già accoglieva il fratello uterino del giovane G. S. e si impegnava, con questo provvedimento, a salvaguardare gli incontri del bambino con il fratello e con il padre. La corte d'appello di Firenze sospendeva comunque il decreto e, con un'ordinanza del novembre 2006 disponeva una consulenza d'ufficio per una valutazione più adeguata della situazione comportamentale. Sennonché, interveniva una segnalazione da parte degli insegnanti del minore e degli assistenti sociali che segnalavano l'estremo disagio della situazione del minore e il comportamento inadeguato del padre, sicché il tribunale revocava, in via provvisoria, la sospensione del provvedimento che era intervenuta, disponendo l'affidamento del minore al responsabile dei servizi sociali del Comune di Firenze e disponendo che, in attesa di una sua collocazione in una famiglia, lo stesso venisse accolto in una struttura. L'ordinanza veniva eseguita il 25 maggio 2007 a cura della polizia municipale che operò in una situazione di totale normalità. Il deposito della consulenza tecnica disposta poneva in evidenza la grave situazione del bambino e poneva delle prescrizioni cui attenersi. L'ordinanza L'ordinanza del 2007 veniva quindi confermata dalla corte d'appello con una serie di provvedimenti che, in via provvisoria, venivano analiticamente previsti nell'interesse del minore e nella prospettiva di favorire comunque gli incontri con il genitore. Per quanto riguarda il successivo aspetto, ossia le specifiche modalità attuate per il prelievo del minore dall'istituto scolastico, il dipartimento per la giustizia minorile ha riferito che l'esecuzione del decreto della corte d'appello è stata curata dal servizio sociale che ha organizzato l'accoglienza del minore presso il "Centro Sicuro" del Comune di Firenze,

Si è ritenuto, in questa occasione, di prelevare il minore durante le ore scolastiche per evitare che potessero esserci interventi reattivi da parte del genitore, che avrebbe potuto anche ostacolare l'esecuzione del provvedimento. Il bambino venne accompagnato nella struttura protetta da persone da lui conosciute, da un'educatrice scolastica, che già costituiva punto di riferimento per il bambino, da un assistente sociale che già da tempo lo seguiva, dalla responsabile e dalla vice responsabile del servizio. L'intervento della Polizia municipale si limitò esclusivamente alla notifica del provvedimento. La stessa Polizia municipale non ebbe alcun contatto con il bambino. Al genitoredel minore veniva comunicato, da parte del responsabile del servizio, la collocazione del bambino nel "Centro Sicuro", spiegando che la sistemazione era provvisoria e che per le caratteristiche del centro non era possibile comunicare l'indirizzo. Peraltro, venivano organizzati gli incontri tra il genitore e il bambino. Il servizio sociale "Centro Sicuro" è struttura protetta il suo indirizzo è segreto nel senso che è conosciuto esclusivamente dagli uffici preposti (uffici del Comune, organi di Polizia, autorità giudiziaria). Si tratta di un istituto di prima accoglienza attivato tramite un protocollo d'intesa tra vari soggetti istituzionali specializzato ad accogliere minori in situazioni di emergenza.

Il Centro possiede tutti i requisiti di affidabilità ed agibilità ed ha l'autorizzazione al funzionamento in base alla documentazione tecnica depositata negli uffici del Comune di Firenze. Il minore, a far data dal 2 luglio, è stato collocato presso una casa famiglia di Forlì. In ottemperanza alle disposizioni della corte d'appello sono stati organizzati incontri tra il padre e il bambino

ma il genitore successivamente produceva una certificazione medica attestante una sua impossibilità a recarsi a Forlì per incontrare il figlio. Tutti gli altri provvedimenti adottati nel decreto dell'autorità giudiziaria sono stati puntualmente Il servizio sociale del Comune di Firenze ha segnalato infine che sarà sua cura reperire altra struttura idonea nel territorio fiorentino, e ciò compatibilmente con il progetto educativo e psico-sociale del minore e con le future determinazioni dell'autorità giudiziaria. In ogni caso, l'inserimento del bambino nella casa famiglia di Forlì è avvenuto in ottemperanza a tutte le disposizioni giudiziarie, prescindendo da valutazioni di tipo economico. Si rappresenta, da ultimo, che durante il periodo di permanenza nel "Centro Sicuro" gli incontri tra il minore e la psicologa che lo seguiva sono stati regolarmente effettuati.

meritevole di ulteriori attenzioni e provvedimenti. La Presidenza, pertanto, si impegna a riprendere le questioni così drammatiche da lei sollevate per ottenere un ulteriore supplemento di conoscenze e di intervento. RAME

previdenza sociale*. Signor Presidente, l'atto ispettivo, presentato dal senatore Sodano, riguarda la situazione aziendale della Fiat Group, con specifico riferimento allo stabilimento di Pomigliano d'Arco ed alle aziende dell'indotto. La Fiat Group, nell'ambito di un piano di riorganizzazione volto a completare l'integrazione dello stabilimento di Pomigliano nel suo sistema produttivo, ha previsto di sospendere l'attività lavorativa, per il periodo dal 7 gennaio al 2 marzo 2008. La società, con riferimento a tutti gli stabilimenti del gruppo, ha individuato, come peraltro evidenziato nell'accordo stipulato in data 22 giugno 2007 tra l'azienda e organizzazioni sindacali nazionali e territoriali FIOM-CGIL, FIRN-CISL, UILM-UIL e FISMIC, un esubero complessivo di circa 1.300 dipendenti. Tra questi, circa 300 sono stati individuati presso il sito produttivo di Pomigliano d'Arco. L'accordo predetto individua i criteri in base ai quali procedere alla collocazione in mobilità dei lavoratori in esubero prevedendo, in particolare, che la messa in mobilità avvenga innanzitutto su base volontaria, valutandosi il possesso dei requisiti di anzianità e di contribuzione utili al pensionamento. Dalle notizie fornite dai responsabili dello stabilimento in questione, alla data del 31 dicembre 2007, risulterebbero collocati in mobilità 296 lavoratori, di cui 221 su base volontaria. Per i restanti 75 dipendenti l'azienda ha proceduto ad inviare le lettere di collocazione in mobilità; tra questi, 56 lavoratori hanno in seguito raggiunto un accordo con l'azienda. Il fermo produttivo dello stabilimento di Pomigliano d'Arco ha determinato, come evidenziato nell'atto ispettivo, conseguenze anche sulle aziende dell'indotto operanti sia all'interno che all'esterno del comprensorio industriale. In particolare, per quanto attiene alle giornate di mancata attività lavorativa nei giorni 10, 11, 12, 18 e 19 dicembre 2007 - causate dal blocco degli autotrasportatori e dallo sciopero proclamato dai dipendenti della DHL Automotive srl operante nel medesimo sito produttivo - l'azienda ha affermato di avere inoltrato all'INPS, in conformità a quanto concordato con le rappresentanze sindacali unitarie dello stabilimento di Pomigliano d'Arco, la richiesta di intervento di trattamento di integrazione salariale ordinario. Con riferimento sempre alla società DHL, per il periodo di fermo dell'attività dal 7 gennaio al 2 marzo 2008, in aderenza a quanto concordato con le organizzazioni sindacali

per un numero massimo di 502 lavoratori. Sulla base delle notizie acquisite, la società DHL, le organizzazioni sindacali territoriali e le rappresentanze sindacali unitarie si sarebbero impegnate ad effettuare, entro il prossimo 28 febbraio, una verifica al fine di esaminare la possibilità di stabilizzare circa 100 lavoratori in precedenza assunti attraverso contratti di somministrazione. Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto, peraltro, che il Gruppo FIAT, con un comunicato del 4 dicembre ultimo scorso, ha deciso di assumere l'impegno di completare l'integrazione dello stabilimento di Pomigliano nel suo sistema produttivo. Tale impegno si realizzerà attraverso un importante piano di investimenti tecnologici da 70 milioni di euro complessivi e un rilevante intervento di formazione dei dipendenti. L'obiettivo è quello di portare lo stabilimento di Pomigliano al livello della migliore concorrenza e creare le condizioni indispensabili per produrre in quella sede i nuovi modelli. In tal modo la società conferma il proprio intendimento di dare prospettive di continuità e sviluppo all'impianto in questione, attraverso interventi sul versante economico ed organizzativo. In conclusione, sono sicuramente in grado di garantire la massima attenzione da parte dell'amministrazione che rappresento in ordine alle situazioni descritte, in considerazione del rilevante impatto che queste hanno sul versante occupazionale e, più in generale, sull'economia del Paese, garantendo, sin d'ora, ogni

il Parlamento e le riforme istituzionali - l'Ufficio interrogazioni, per l'esattezza - ha assicurato che seguirà la vicenda da lei sollevata presso gli uffici competenti del Ministero della giustizia. Lo seguiremo e sarà mia cura tenerla informata, ma immagino che sarà informata lei stessa

era già una prima reazione, così aspra, da parte dell'azienda, con il licenziamento di sette lavoratori, ciò creava qualche dubbio anche sulla bontà dei buoni propositi dell'accordo firmato nel dicembre 2007.

venga presentato e rispettato il Piano industriale aziendale, che garantisca appunto quei livelli occupazionali cui faceva riferimento il sottosegretario Montagnino nella parte finale della sua risposta.

al rinnovo e all'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia. Inoltre, per finanziare anche progetti di potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, la stessa finanziaria ha istituito un Fondo per la legalità, nel cui ambito reperire ulteriori risorse, alimentato dalle somme dei beni immobili confiscati alla mafia, in applicazione della legge n. 575 del 1965. In relazione alla situazione delle autovetture in dotazione alla Questura di Vicenza e al Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa, risponde al vero che la dotazione dei mezzi presentava criticità alla data del 10 novembre 2006, quando è stata effettuata la rapina ai danni dell'istituto di credito Deutsche Bank, sito in Piazzale Giusti a Vicenza. che le risorse finanziarie assegnate al Ministero dell'interno per la manutenzione ed il rinnovo dei mezzi hanno registrato, nel periodo 2004-2007, un andamento tendenzialmente decrescente. A fronte di tale situazione, l'amministrazione dell'Interno si è prontamente attivata con un'attenta opera di razionalizzazione della spesa, dando luogo ad una graduale sostituzione dei veicoli destinati al controllo del territorio e all'adozione di pacchetti di manutenzione, finalizzati a contenere la spesa occorrente per gli interventi di riparazione dei mezzi. Ciò ha consentito, già dal mese di gennaio dello scorso anno, di ripianare, almeno parzialmente, le carenze della Questura di Vicenza, con l'assegnazione di un'autovettura Alfa Romeo 147, con colori di serie,

risulta sufficiente rispetto alle necessità del territorio provinciale e non presenta evidenze negative. Le vetture a disposizione della Questura di Vicenza e del Commissariato di Bassano del Grappa sono infatti 44, anche se due di queste in attesa di riparazione. Per quanto riguarda la situazione delle risorse umane, cui fa riferimento l'interrogante, preciso che negli uffici di Vicenza e Bassano del Grappa prestano servizio 352 appartenenti ai ruoli operativi della Polizia rispetto ad un organico di 288 unità. Contribuiscono alla funzionalità delle due strutture 38 operatori dei ruoli tecnici e 44 dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno; inoltre, di recente sono stati assegnati in via temporanea per le esigenze dell'Ufficio immigrazione due agenti ausiliari trattenuti provenienti dal 63° e dal 64° corso e altre quattro unità saranno assegnate alla Questura entro la fine del primo semestre del corrente anno.

L'interrogazione, come lei ha ricordato, prendeva spunto da un fatto di cronaca clamoroso: il locale quotidiano aveva riportato la notizia che i poliziotti della squadra mobile del posto, il giorno 10 novembre 2006, erano dovuti uscire a piedi per sventare una rapina presso l'agenzia della Deutsche Bank di Vicenza a causa della mancanza di automezzi a disposizione, che erano tutti in riparazione. Peraltro, io stesso, in una precedente interrogazione del 7 novembre 2006, che nel frattempo è rimasta priva di riscontro, avevo denunciato proprio questa penosa situazione del parco macchine della Questura di Vicenza, che era dotato soltanto di Fiat Marea, che avevano oltre 200.000 chilometri ciascuna, che spesso non non erano utilizzabili e che anzi talvolta erano fuori norma secondo la motorizzazione. Oggi lei, onorevole Sottosegretario, viene a dirci che la situazione è migliorata in quanto nel frattempo sono arrivate in dotazione alle volanti della squadra mobile di Vicenza dei nuovi mezzi. Di questo prendiamo atto, anche se nel frattempo rimane inadeguata la dotazione sia delle auto civetta, sia delle auto utilizzate per le scorte. rispetto al novembre 2006, quando i poliziotti di Vicenza dovevano rincorrere i rapinatori a piedi, la situazione è migliorata, ma ci mancherebbe altro! Peraltro, le Alfa Romeo 159 che lei ha citato, secondo quanto ci riferiscono gli operatori del settore, non sono proprio il massimo per le esigenze operative: sono delle autovetture *diesel* e in talune situazioni hanno dimostrato di non avere l'agilità necessaria per lo svolgimento delle funzioni alle quali sono assegnate. In effetti, nonostante l'arrivo di questi automezzi, nel complesso la situazione operativa della Questura di Vicenza rimane allarmante; pensi, onorevole Sottosegretario, che poche settimane fa, solo a seguito dell'intervento dell'Associazione delle piccole e medie imprese della Provincia di Vicenza, su segnalazione del sindacato di polizia, la Polizia postale - che,

dell'Associazione delle piccole e medie imprese della Provincia di Vicenza, la polizia postale non avrebbe potuto svolgere il proprio lavoro. Purtroppo, onorevole Sottosegretario, anche nella nostra Provincia, a seguito di un'immigrazione spesso incontrollata, gli indici di criminalità sono in considerevole aumento: rapine, spaccio di sostanze stupefacenti, prostituzione, immigrazione clandestina, difficoltà nell'identificazione degli stranieri, aggravata dal sempre più diffuso fenomeno del falso documentale, ma anche il rischio terrorismo, legato alla realizzazione della nuova base americana presso l'aeroporto «Dal Molin», imporrebbero un controllo del territorio sempre più capillare. In effetti, non bastano a garantire la sicurezza dei cittadini le due volanti che ogni notte operano sull'intero territorio provinciale. Da pochi giorni si è insediato a Vicenza il nuovo questore, il dottor Sarlo, l'occasione ci è utile per fargli l'augurio di un buon lavoro.

istituzionali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, prima dì rispondere all'interrogazione del senatore Paravia, desidero ribadire, a nome del Governo e mio personale, la piena solidarietà nei confronti di tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, che quotidianamente, rischiando la vita, garantiscono la sicurezza dei cittadini. E' il caso dell'ispettore superiore, sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, Filippo Raciti che, come testimonia la motivazione del conferimento della medaglia d'oro al valor civile, il 2 febbraio 2007 - cito testualmente - «con spiccata professionalità, non comune determinazione operativa e consapevole sprezzo del pericolo, si prodigava nel fronteggiare e respingere un gruppo di facinorosi tifosi catanesi, rimanendo mortalmente ferito nei corso dei violentissimi scontri». La credibilità delle istituzioni e dello Stato nella coscienza dei cittadini pretende che a tali riconoscimenti seguano misure tempestive anche di carattere economico alle famiglie di tali eroi così drammaticamente e duramente colpite e, nel caso di cui ci stiamo occupando, a sostegno dalla vedova Raciti, signora Marisa Grasso e dei figli minori, Alessio e Fabiana. Informo il Senato che il Ministero dell'interno - che si è costituito parte civile nei procedimenti penali instaurati per i fatti accaduti ha corrisposto, a decorrere dal 1° marzo 2007, la pensione ordinaria indiretta (per un importo netto mensile di circa 1.400 euro) e, dal successivo mese di luglio, ma con decorrenza sempre dal 1° marzo, la liquidazione del trattamento pensionistico speciale (per un importo netto mensile di circa 2.417 euro). Quest'ultimo importo è commisurato agli emolumenti attribuiti al personale in servizio con qualifica superiore a quella di Raciti alla data del decesso e sarà aggiornato sulla base dei relativi aumenti di stipendio. Questo perché, con decorrenza del 2 febbraio scorso, l'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti è stato promosso, per merito straordinario, alla qualifica di ispettore superiore e i suoi eredi avranno quindi diritto a tale trattamento pensionistico. Con mandato del 26 febbraio 2007, la sede dell'INPDAP di Catania ha corrisposto alla signora Grasso, vedova Raciti, l'indennità di buonuscita, calcolata in base all'anzianità previdenziale maturata dal marito (per un importo netto di circa 35.600 euro). Con decreto ministeriale del 29 maggio 2007, l'Amministrazione dell'interno ha inoltre provveduto a liquidare alla signora Grasso l'equo indennizzo di prima categoria (pari a circa 39.500 euro netti). Tutti i benefìci di natura previdenziale previsti dalla vigente normativa sono stati corrisposti nella piena osservanza dei termini del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241 del 1990. Con pari tempestività sono state completate le procedure finalizzate alla concessione delle speciali elargizioni spettanti, in base alla normativa vigente, alla famiglia dell'ispettore superiore Filippo Raciti, quale vittima del dovere. Infatti, il 13 novembre 2007 è stato adottato, in favore della vedova e dei due figli minori, il decreto per la concessione della speciale elargizione in misura massima, rivalutata secondo l'indice ISTAT (circa 220.700 euro). II successivo 14 novembre è stato emanato anche il provvedimento relativo all'attribuzione dell'assegno vitalizio mensile che spetta non solo alla signora Grasso, ma anche a ciascuno dei due figli. Detto importo, non reversibile, è esente dall'IRPEF ed è soggetto a perequazione automatica. Le somme destinate ai minori verranno elargite non appena perverrà al Ministero dell'interno, che ne ha già sollecitato il rilascio, l'atto con cui il giudice tutelare dispone l'impiego degli importi. Oltre ai benefìci di natura economica, le vigenti disposizioni prevedono l'assunzione diretta nelle qualifiche iniziali di agente o di operatore tecnico della Polizia di Stato, in favore dei componenti del nucleo familiare, di un operatore di Polizia vittima del dovere. Ciò a condizione che i beneficiari ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti necessari. Poiché la signora Grasso non ha finora presentato alcuna richiesta di assunzione, detto beneficio potrà eventualmente essere fruito dai due figli al raggiungimento della maggiore età. Da quanto sopra esposto, emerge con evidenza che il Ministero dell'interno ha espletato ogni adempimento a favore del nucleo familiare dell'ispettore superiore Filippo Raciti. Assicuro che uguale impegno viene profuso per l'espletamento di tutte le procedure amministrative volte all'erogazione dei benefìci di cui alla normativa menzionata dagli onorevoli interroganti. Da tempo è in atto una progressiva estensione dei benefìci già previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha autorizzato la spessa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2006. Tenuto conto della limitatezza degli stanziamenti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 7 luglio 2006 ha previsto la formazione di una graduatoria unica nazionale di tutte le posizioni tutelate, secondo l'ordine cronologico. Ricordo che lo stesso regolamento differenzia i benefìci economici secondo l'entità del danno e riserva la somma di 500.000 II Governo, tenuto conto dell'importanza di assicurare prontamente

per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009, per le speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti e alle vittime della criminalità organizzata. Inoltre, la legge finanziaria del 2008 riconosce, a decorrere dal corrente anno, alle vittime della criminalità organizzata e del dovere, ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni, nonché ai loro familiari superstiti, i benefìci economici delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Per quanto riguarda infine i procedimenti pendenti in attesa di risarcimento, preciso che al momento, su un totale di 938 richieste, ne sono state definite 532 (cioè il 57 per cento) e sono in istruttoria 406 casi. Relativamente a questo ultimo dato, va precisato che dal 15 ottobre ad oggi sono pervenute 200 richieste relative alla legge n. 266 del 2005 e 145 in applicazione di altre normative sulle vittime del dovere. II Governo si sta adoperando anche per semplificare i procedimenti amministrativi per la concessione di tali benefici. Ricordo che sulla base dell'articolo 3 della delega prevista dalla legge di semplificazione per l'anno 2005, il Ministero dell'interno sta predisponendo uno schema di provvedimento normativo, da sottoporre all'esame di un apposito tavolo tecnico interministeriale, già istituito,

la tempestività con cui sarebbero stati corrisposti alla vedova Raciti tutti i suoi diritti, per sé e per i suoi figlioli. La prego però vivamente, senza costringermi a ripresentare un'ulteriore interrogazione,

di Stato per l'interno*. Il prefetto di Frosinone e le autorità provinciali di pubblica sicurezza ci riferiscono che il 13 dicembre

Nell'imminenza della cerimonia, il comandante della locale Polizia municipale, unitamente al proprio personale, ha invitato i dimostranti a rimuovere manifesti e striscioni, nonché a desistere dalla divulgazione di volantini, quanto attività ritenute in violazione del divieto posto da vigenti ordinanze comunali in materia di decoro urbano. Ne è scaturita una vivace protesta nel corso della quale uno striscione rimaneva danneggiato, mentre l'altro veniva successivamente rimosso dagli stessi manifestanti. Dagli elementi acquisiti emerge che il citato episodio non ha comunque impedito la prosecuzione dell'iniziativa. Tuttavia, il giorno seguente il presidente del circolo di Alleanza Nazionale ha trasmesso alla procura della Repubblica di Cassino, nonché al Ministero dell'interno, al prefetto di Frosinone e ai Carabinieri di Isola del Liri, una denuncia nella quale, richiamando quanto avvenuto, ha contestato nella condotta dei vigili urbani gli estremi dell'abuso d'ufficio e della violenza privata. Sugli stessi fatti anche il predetto ufficio della Polizia municipale ha fornito la propria versione, inviando all'autorità giudiziaria una nota informativa allo scopo di chiarire le fasi della vicenda e consentire la valutazione di eventuali ipotesi di reato a carico del promotore dell'iniziativa e di altri manifestanti. Secondo quanto riferito dal Ministero della giustizia, a seguito dell'esposto inoltrato dal presidente del circolo di Alleanza Nazionale, il procuratore della Repubblica di Cassino ha avviato un apposito procedimento penale, le cui indagini, tuttora in corso, sono state delegate al locale Comando stazione dei Carabinieri. Pur in attesa delle determinazioni di competenza dell'autorità giudiziaria, sottolineo, secondo quanto riferito dalla prefettura dì Frosinone, che presso il Comune di Isola del Liri, al di là delle contrapposizioni (anche vivaci) che caratterizzano i locali rapporti tra le opposte componenti della civica amministrazione, non sussistono significative condizioni di tensione e turbamento atte a pregiudicare la serenità e la convivenza di tutte le forze politiche. Assicuro, comunque, che il Ministero dell'interno, attraverso la predetta prefettura e le altre autorità provinciali di

la signora Sottosegretario per la risposta all'interrogazione, che purtroppo non soddisfa la richiesta iniziale,

presa come un silenzio‑assenso da parte dell'amministrazione comunale del Comune di Isola del Liri. Del resto, è molto discutibile il fatto che vi siano delle ordinanze da parte del sindaco, o comunque delle autorità comunali di quel paese, in materia di decoro urbano. Qui è stato spostato l'asse del tema posto dalla mia interrogazione. D'altra parte, se vi fosse stata una qualsiasi deturpazione non avremmo avuto la possibilità di leggere, e quindi di sentire anche dal Sottosegretario, che un manifesto era stato strappato. Quindi, si è trattato di una manifestazione civilissima, di contestazione, da parte dell'opposizione, con i rappresentanti di Alleanza nazionale, dell'UDC e di Forza Italia. Non è vero che in quel Comune c'è un clima sereno, signora Sottosegretario: è esattamente il contrario. C'è un clima abbastanza teso e di contrasto, soprattutto legato, per notizie che mi constano direttamente e che quotidianamente sono anche sulla stampa locale, ad una scarsa disponibilità da parte del sindaco e dell'amministrazione a voler avere un rapporto ed un dialogo con le opposizioni e a permettere alle stesse di esprimersi nel modo più libero e compiuto. Del resto, questi fatti stanno a documentare la volontà da parte degli amministratori, sia pure tramite i vigili urbani, di impedire una manifestazione che, alla fine, non era nient'altro che una protesta protesta civile nei confronti di un'iniziativa che l'opposizione non riteneva valida e, comunque, ha argomentato anche su questo. Mi auguro che vi possa essere maggiore attenzione, ma soprattutto che anche dall'iniziativa del procuratore della Repubblica di Cassino, così come ha riferito la signora Sottosegretario, possa venire fuori il dato che, di fatto, non è stato permesso a dei cittadini, che lo avevano richiesto formalmente, di manifestare le proprie intenzioni e, quindi, le proprie opinioni, e pertanto gli stessi sono stati conculcati in quelle libertà fondamentali che la nostra Costituzione garantisce.

È del tutto evidente che ho sbagliato, nel senso che la mia intenzione era di votare contro; purtroppo, il mio voto a favore è stato determinante nell'approvare il dispositivo della risoluzione.

una nuova finestra"). Colleghi, comunico di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio dei ministri la seguente lettera: Onorevole Presidente, Informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dal sen. dott. Clemente MASTELLA, senatore delle Repubblica, dalla carica di Ministro della giustizia.

del Presidente del Consiglio dei ministri relativa alle dimissioni del Ministro della giustizia. Potranno pertanto intervenire un senatore per Gruppo per dieci minuti e i rappresentanti del Gruppo Misto per complessivi quindici minuti. Non sono previste votazioni. La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre stabilito che la Relazione del Ministro della giustizia sullo stato della giustizia e conseguente dibattito, secondo le modalità già definite dalla precedente Conferenza dei Capigruppo, si svolgeranno nella seduta antimeridiana di giovedì 24 gennaio, a partire dalle ore 9 e fino alla conclusione delle votazioni. La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi nella giornata di martedì 22 gennaio per la definizione del calendario successivo.

sono qui oggi in quest'Aula del Senato per comunicarvi l'orientamento maturato dal Governo a seguito degli avvenimenti della giornata di ieri. Chiamato ieri mattina in Parlamento a illustrare le linee della politica del Governo in tema di giustizia, il Ministro Guardasigilli ha affrontato la situazione creatasi con l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti In quello che è stato il discorso più difficile e sofferto della sua lunga vita politica, Clemente Mastella ha parlato da uomo offeso nel proprio onore e colpito negli affetti più cari. A lui come Ministro, come collega, come politico e come amico, voglio esprimere di fronte a voi la mia profonda solidarietà. Il Ministro della giustizia non ha esitato a far prevalere le ragioni dell'onore e della dignità sua personale e della sua famiglia su tutte le altre motivazioni che avrebbero potuto, come politico, suggerirgli comportamenti diversi. Non ha esitato e perciò ha presentato le proprie dimissioni. ha scelto di presentare le proprie dimissioni di fronte al Parlamento testimoniando, anche in questo modo, una sensibilità istituzionale che, nella nostra società delle comunicazioni ed in una stagione nella quale la politica troppo spesso si fa spettacolo, si va facendo sempre più rara. Tutti ieri hanno colto l'emozione e la commozione con le quali ha parlato il ministro Mastella. La sincerità dei sentimenti che lo muovevano e la nobiltà della scelta di rimettere il proprio mandato si sono riflesse nella reazione dell'Assemblea di Montecitorio che, con una coralità che ha travalicato gli steccati che dividono gli opposti schieramenti politici, ha espresso il proprio pieno apprezzamento al Ministro. Questa medesima valutazione, con l'apprezzamento e la condivisione del lavoro da lui fatto sin dall'avvio del Governo alla guida del Dicastero della giustizia, mi hanno indotto, nella tarda mattinata di ieri, a respingere le dimissioni del ministro Mastella e a chiedere a lui di continuare la propria opera per assicurare un'amministrazione della giustizia sempre più efficiente e all'altezza delle esigenze e delle aspettative della società italiana. Alla mia decisione di respingere le sue dimissioni, il ministro Mastella ha risposto chiedendo una pausa di riflessione che gli permettesse, innanzitutto, di raccogliersi con la sua famiglia. Ieri sera e, di nuovo, questa mattina Mastella mi ha, però, confermato che la sua determinazione non era mutata. L'estendersi, sempre nella giornata di ieri, dei provvedimenti della magistratura direttamente alla sua persona non aveva fatto che rafforzare le ragioni di una decisione che egli aveva già pienamente assunto. A Clemente Mastella va - ve lo ripeto ancora una volta - la mia solidarietà piena e affettuosa, ed analoga solidarietà voglio esprimere al suo partito, ai Popolari-Udeur, sul cui appoggio il Governo ha contato in passato e conta per il futuro. Ho parlato prima di preoccupazione per un'azione di Governo che deve proseguire senza interruzioni e senza perdite di velocità. Questa preoccupazione l'ha avvertita e riconosciuta il senatore Mastella nel determinarsi a presentare e poi a confermare le proprie dimissioni. Come Presidente del Consiglio l'ho avvertita io stesso e l'ho fatta mia. È per questo che ho proposto al Capo dello Stato di assumere io stesso, *ad interim,* la responsabilità di Ministro della giustizia. In un incontro, nel primo pomeriggio, al Palazzo del Quirinale, il presidente Napolitano ha accettato questa mia proposta ed ha firmato il decreto della mia nomina a Ministro della giustizia. La scelta di caricarmi personalmente, in una prospettiva limitata nel tempo, di questa responsabilità è e vuole dichiaratamente essere il segnale di un'attesa. L'attesa, cioè, che dalla magistratura possa, nei tempi più rapidi possibili, giungere un chiarimento forte che consenta al senatore Mastella di riprendere, con ritrovata e piena autorità, il suo posto di Ministro della giustizia. Le scelte che vi ho ora illustrato, e della cui maturazione ho costantemente tenuto informato il Capo dello Stato, assicurano ed assicureranno al Governo un'intatta capacità di conduzione della politica giudiziaria. Egualmente esse assicurano ed assicureranno al Governo la solidità e la continuità dell'appoggio politico della propria maggioranza. La giornata di ieri era dedicata, secondo il calendario della Camera dei deputati, al dibattito sullo stato della giustizia. obiettivo era concentrata l'ampia relazione che il Ministro Guardasigilli aveva preparato e che gli avvenimenti della giornata lo hanno costretto a consegnare per iscritto, senza che su di essa si potesse poi svolgere il previsto e dovuto dibattito. Nella mia nuova funzione di Ministro della giustizia assicurerò che questo dibattito possa avvenire, nei tempi decisi dal Parlamento, in forma esaustiva, a partire proprio dalla relazione che è stata che è stata consegnata ieri alla Camera. Potranno essere così compiutamente esaminati e discussi tanto il bilancio consuntivo quanto le prospettive dell'azione di Governo e le prospettive della giustizia nel nostro Paese. Come Ministro Guardasigilli mi impegno, sin d'ora, a proseguire la politica di trasparenza, di rispetto dell'indipendenza della magistratura e della tutela dei diritti delle persone, a partire dalla presunzione di innocenza del cittadino indagato, che ha caratterizzato l'attività di questi primi venti mesi di Governo e che è il presupposto di ogni sistema democratico. Sempre nel corso della prossima settimana, l'inaugurazione dell'anno giudiziario mi offrirà un'ulteriore occasione per illustrare le linee guida dell'azione che il Governo intende seguire per dare agli italiani quella giustizia sempre più giusta, rapida ed efficiente a cui essi hanno diritto.

e in tal senso, a maggior ragione, noi tutti dobbiamo interpretarle al meglio, cioè con senso di responsabilità, rispetto istituzionale e dimensione del ruolo che ciascuno di noi riveste in quest'Aula. Pertanto, in questo momento, in cui ci stiamo confrontando in merito alle dimissioni del ministro della giustizia, Clemente Mastella, non dobbiamo perdere di vista quelle che a nostro avviso, ad avviso dei senatori di Italia dei Valori, sono due delle principali architravi che sostengono la nostra democrazia: il rispetto per le istituzioni, per tutte le istituzioni, ed il rispetto dei cittadini per il consenso che ci hanno dato e quindi per la sovranità popolare che in questo momento, da questi scranni, rappresentiamo. Nel far ciò, signor Presidente, non possiamo innanzitutto non partire proprio dal comportamento del senatore Mastella, del quale abbiamo apprezzato in quest'anno e mezzo, la fatica ed il lavoro ad un Dicastero assai difficile, complesso, articolato; l'impegno verso le istituzioni e il rispetto - sempre dimostrato - per quest'Aula e per il Paese. Proprio per questi motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo vicini al dramma umano che sta vivendo il senatore Mastella. Un dramma - ed uso queste parole proprio in ragione di quanto ieri ed oggi ha avuto modo lui stesso di dire nel nostro Parlamento - che nasce dal sentire gli affetti più cari in una situazione di difficoltà. Capiamo il dramma, la difficoltà, ed in questo la nostra solidarietà è massima. Alla solidarietà umana aggiungiamo anche quel tipo di solidarietà che nasce dal rispetto per la scelta - che per noi non può che essere evidentemente obbligata - delle dimissioni da Guardasigilli che egli ha voluto rassegnare. Dimissioni per noi obbligate. Tuttavia, signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione di oggi non può fermarsi qui. Essa deve affrontare con chiarezza - nel rispetto della separazione dei poteri dello Stato e delle nostre istituzioni, insomma della nostra democrazia - il fatto che le dichiarazioni che il senatore Mastella e l'uso che ha voluto riservare, attraverso la scelta delle parole, alla magistratura e ai magistrati sono stati inopportuni. Prendiamo atto comunque che oggi il ministro Mastella, in una conferenza stampa, ha fatto delle importanti dichiarazioni a favore del ruolo della magistratura, giustificando il suo intervento di ieri un po' duro, perché segnato dall'emozione del momento. Quelle parole, ancor di più perché pronunciate dal Ministro della giustizia, hanno determinato un inopportuno cortocircuito tra due princìpi previsti dalla Carta costituzionale che non devono essere mai posti in conflitto: piena indipendenza dell'autonomia della magistratura, da una parte, e presunzione di non colpevolezza sino alla sentenza passata in giudicato, dall'altra. A proposito dei provvedimenti giudiziari, sicuramente il tempo chiarirà ogni aspetto di questa vicenda processuale. Signor Presidente del Consiglio, noi senatori dell'Italia dei Valori, come ha già dichiarato il nostro presidente Antonio Di Pietro, auspichiamo la nomina nel breve periodo di un Ministro che possa, a tempo pieno, dedicarsi alle questioni della giustizia. Insomma, signor Presidente, ci auguriamo che il suo interinato duri il meno possibile.

di fronte ad una vicenda di malaffare che coinvolge un Ministro della sua coalizione e un partito della sua maggioranza. Ella ha tentato invano di resistere all'ondata di fango che vi è piovuta addosso; ha persino proposto al senatore Mastella di restare al proprio posto, ma questi le ha risposto di no, e non per sensibilità istituzionale (come si continua provocatoriamente e ipocritamente a ripetere), ma molto più semplicemente perché ha detto di avere paura. Signor Presidente del Consiglio, lei non ha paura nel momento in cui assume l'*interim* della giustizia? Oppure considererà un vile chi si dimette, come ha fatto il ministro Mastella? Signor Presidente del Consiglio, c'è anche qualche altra domanda che vorrei porle, alle quali sono certo non darà risposta, come recentemente ha cominciato a fare persino con i giornalisti. Il Ministro della giustizia - ha ragione il collega Giambrone è l'unico titolare di funzioni di governo citato nella Costituzione assieme al Presidente del Consiglio dei ministri. In questo momento, lei assume, con l'*interim*, un potere costituzionalmente rilevantissimo, sul quale non so se esistano precedenti. È sicuro di non dover sollecitare un voto di fiducia per spiegare se intende proseguire lungo la linea descritta oralmente ieri alla Camera dal suo predecessore di via Arenula e su come eserciterà le funzioni di Ministro della giustizia, secondo quanto allo stesso viene delegato dalla Costituzione? La prego di ascoltarmi, signor Presidente del Consiglio, perché di queste domande è piena la Nazione. Intende promuovere ancora l'azione disciplinare contro il pubblico ministero De Magistris? Sarà più o meno sereno di Mastella quando dovrà inviare ispettori presso gli uffici giudiziari che indagano sulla sua persona? Vale la pena di esporre il Presidente del Consiglio, e soprattutto il Paese, al rischio di nuove figuracce su un tema che vede la politica scattare come una molla quando si tocca un uomo politico e mai quando capita ad un cittadino? Le rivolgo la prima interrogazione orale, se mi permette, signor Ministro della giustizia; quello che denuncio è un fatto gravissimo. Apprendo da un'agenzia di stampa che il senatore Mastella ha appena fatto visita ai numerosi esponenti del suo partito agli arresti domiciliari. Da nuovo Guardasigilli le chiedo di verificare se è vero, perché questo non può farlo neppure un parlamentare, figuriamoci un coimputato. I parlamentari possono fare visite nelle carceri per verificare le condizioni dei detenuti, non nelle loro case dove stanno agli arresti domiciliari: è vietato dalla legge! Non vorrei che fosse un atto di cinismo per far arrestare le persone che stanno agli arresti domiciliari - perché questo dovranno fare i magistrati - e innescare una nuova campagna di vittimismo. Mi rifiuto di pensare che possa esserci un magistrato che autorizza la visita di un coimputato! Quello che è accaduto questo pomeriggio, se è vero, è davvero di inaudita gravità! Signor Presidente del Consiglio, lei avrebbe molte ragioni per aver paura di assumere l'incarico, soprattutto se dovesse continuare nella stessa linea seguita dal suo predecessore, persino in questi momenti. Credo che l'Italia abbia bisogno di rispetto. Credo che l'Italia aspetti che anche lei se ne vada: sarà la prima volta che guadagnerà la gratitudine dell'intero popolo italiano!

Signor Presidente del Consiglio, la scelta di assumere l'*interim* della giustizia è quella più logica e più corretta, e noi dell'Unione Democratica la condividiamo totalmente; così come comprendiamo la scelta di un *interim* che rispetti i problemi del ministro Mastella aspettandone la soluzione. Bene ha fatto, poi, il senatore Mastella a confermare le sue pronte dimissioni, scegliendo di difendersi a mani libere nel processo e non dal processo. A tal proposito, gli auguriamo di poter vedere quanto prima acclarata la sua estraneità, rinnovando insieme a lui la fiducia nella funzione che svolge la magistratura nel suo complesso. Abbiamo l'obbligo, però, di non nasconderci che un problema esiste da tempo rispetto alle misure cautelari personali che a volte vengono con troppa leggerezza disposte. Mastella ha parlato di "frange estremiste" e di "pacchetto di mischia", ma, superando le definizioni, condivisibili o meno, dobbiamo riconoscere che è ormai indifferibile un intervento modificativo che eviti o limiti eventuali arbitrii perché ogni correzione postuma non potrà mai restituire quello che un arresto affrettato ha tolto. E non dobbiamo farlo perché qualche personaggio illustre che può occasionalmente incorrere in tali anomali ce lo chiede, ma per i tanti cittadini senza volto che difficilmente potranno rappresentare pubblicamente i loro drammi. È allora giunto il momento di pensare ad un nuovo sistema cautelare che preveda, prima, un collegio che decide e, poi, un organismo monocratico che controlla e non l'opposto, come purtroppo accade oggi. Per preservare poi l'autonomia e l'indipendenza dalla magistratura è necessario rafforzare l'effettività della potestà di autotutela, separando nel CSM la funzione disciplinare da tutte le altre. Come vede, Neoguardasigilli, due proposte specifiche sulle quali ci aspettiamo una risposta concreta e puntuale nel corso del prossimo dibattito sulla giustizia. Non voglio però sottrarmi ad una valutazione personale e specifica sulla vicenda. Non sembra raffigurabile alcun illecito penalmente rilevante nel pretendere di poter indicare un assessore o un Ministro. Esiste invece un problema etico che dev'essere affrontato relativamente alla gestione politica della Regione Campania e forse dell'intero Paese. Questo grave problema, a mio avviso, però essere affrontato nelle Aule parlamentari (perché il giudice naturale rispetto a questo problema è il popolo) e non nelle aule di giustizia. C'è poi, signor Presidente del Consiglio, una questione squisitamente politica che le rappresento. Anche in un momento delicato come questo abbiamo dovuto, purtroppo, registrare che esiste di fatto una forte intesa fra i due maggiori partiti che siedono in Parlamento: il Partito Democratico e Forza Italia. Pochi giorni fa, in una riunione di maggioranza, un importante esponente del Partito Democratico ci ha notificato che per la riforma elettorale non esiste uno schieramento precostituito da tutelare, ma la maggioranza dev'essere ricercata in Commissione o in Aula, operando un chiaro riferimento a Forza Italia. Ci è stato notificato, signor Presidente del Consiglio, un avviso di maggioranze variabili, che poche ore fa si è puntualmente materializzato in quest'Aula. Infatti, nella tarda mattinata di oggi, l'assoluta mancanza di una scelta condivisa in una materia delicata come quella relativa alla gestione dei rifiuti in Campania avrebbe potuto determinare la mancata approvazione della proposta di risoluzione del Partito Democratico (non sottoscritta da circa dieci senatori della maggioranza)

condividiamo pienamente, onorevole Prodi, la sua informativa sulle dimissioni del ministro Mastella. Crediamo che abbia operato bene, che il Governo abbia fatto bene e che lei abbia deciso bene di venire qui in Parlamento per rendere queste dichiarazioni. Contemporaneamente, abbiamo apprezzato l'atto del ministro Mastella compiuto ieri alla Camera dei deputati e abbiamo dato al ministro ministro Mastella la nostra solidarietà, che ribadiamo qui oggi. Oggi sappiamo più di ieri delle motivazioni che hanno indotto la procura di Santa Maria Capua Vetere ad assumere le iniziative che ha assunto nei confronti del ministro Mastella e di altri esponenti dell'Udeur della Campania. Per quanto è dato a noi socialisti sapere, manifestiamo molte riserve sulla fondatezza di quella iniziativa. La questione che stiamo affrontando, signor Presidente del Consiglio, come lei ha già accennato, è estremamente delicata: non riguarda solo la vicenda di un Ministro, ma ripropone il tema dei poteri dello Stato e, più precisamente, dei rapporti tra essi e, ancora più specificatamente, tra politica e giustizia, tra magistratura, Parlamento e Governo. Sediamo qui, in questi banchi, signor Presidente, onorevoli colleghi, non perché chiediamo o abbiamo diritto ad alcun salvacondotto rispetto all'azione della magistratura, quando essa lo ritiene opportuno. Le garanzie che pretendiamo siano difese sono quelle previste dalla Costituzione repubblicana, a tutela non delle nostre persone, ma di ciò che rappresentiamo nel nostro ordinamento democratico. Ieri, un nostro autorevole collega ha detto che per emettere una misura cautelare ci vogliono elementi gravi (è il senatore D'Ambrosio che ha rilasciato quest'affermazione); aggiungo che dare notizia alla stampa da parte della magistratura, prima in senso scritto (mi riferisco alle intercettazioni) e poi addirittura a voce (in audio), è un atto di malcostume politico, morale e istituzionale. E che cos'è aprire un'inchiesta, dopo che si è lavorato per mesi su intercettazioni di molte persone, emettendo - com'è stato fatto ieri - un provvedimento di custodia cautelare, per poi comunicare che, però, non essendo per esso competenti, competenti, si trasmettono gli atti ad un'altra procura? Cos'è questo, se non un atto - almeno - di disinvoltura istituzionale? Nella questione delle intercettazioni, signor Presidente si individua spesso una violazione della *privacy* per centinaia di migliaia di cittadini italiani ignari: si rendono pubbliche in scritto e in voce. Non vi è in noi alcun desiderio di aprire inutili polemiche: un uomo pubblico, se sbaglia, deve pagare. Ieri, il direttore di un importante giornale, in una trasmissione televisiva, che la politica non deve dare l'impressione di chiudersi in se stessa in un'autodifesa. Affermazione del tutto condivisibile; qui, però, mi domando se un parlamentare ed un uomo politico abbia diritto di difendersi, solo con la legge e attraverso la legge, rispetto ad accuse che ritiene infondate. Signor Presidente del Consiglio, è nostro convincimento che l'obiettivo delle grandi forze politiche democratiche di questo Paese, anche di fronte ai passaggi cruciali che ci stanno davanti, dovrebbe essere quello di unire l'Italia, l'Italia, in valori condivisi, attorno alle sue istituzioni, democratiche e repubblicane. La democrazia, signor Presidente del Senato, è un equilibrio dei poteri in rapporto con la società: se lo si incrina o lo si spezza, si spezza quell'equilibrio che ci ci fa dire che nei Parlamenti risiede la rappresentanza di un Paese, non altrove, così come la sovranità popolare appartiene al popolo e a nessun altro. Allora, signor Presidente del Consiglio, anche in relazione alle polemiche di queste ore e di questi momenti (ho appreso le dichiarazioni rese, in particolare, dal ministro Di Pietro nei confronti dell'Udeur e dell'onorevole Mastella), vedo la necessità che il Governo compia un attento e coraggioso esame nell'attuazione del programma di legislatura. che affronti con responsabilità, trasparenza e determinazione, signor Presidente del Consiglio, quei problemi politici non risolti che abbiamo di fronte. Occorre un chiarimento vero nella maggioranza, teso a rafforzare l'azione del Governo e a riprendere un cammino e un confronto più aperto in Parlamento per le riforme di cui l'Italia ha bisogno. Non vi è dietro di noi, cioè dietro la politica, una salvifica società civile, ma una società inquieta, non serena, chiusa, non aperta. Ma l'Italia - pensiamo - ha le forze e le energie per guardare avanti, a condizione che riusciamo a darle speranza. *(Applausi dai

Signor Presidente del Consiglio, colleghi senatori, non vorrei replicare al Senato argomenti che il Presidente del Consiglio ha già ascoltato dal nostro Gruppo alla Camera, perché Pomicino gli ha rappresentato, in telepatia con quello che ha detto il senatore Angius, il nesso profondo che c'è tra la vicenda che attraversiamo e la crisi della rappresentanza politica che dobbiamo mettere tutti e tutta intera sulle nostre spalle. Signor Presidente del Consiglio, come sempre accade a chi, pur con qualche distanza temporale da lei, avanza sulla strada della maturità, vengono in questi momenti sempre i ricordi più lontani. Io, quindi, che ho osservato il ministro Mastella per tanti decenni di protagonismo politico (più marcato, in verità, nella seconda Repubblica anziché nella prima), nella solidarietà e nel dolore sincero, non retorico, con cui seguo questa vicenda emotiva e politica, mi sono ritrovato a ricordare alcuni brani della vita di Mastella, i più lontani, ed in particolare uno, che risale ad un'epoca che il presidente Prodi ricorda bene, perché fu anche il suo esordio governativo, gli anni della solidarietà nazionale. Ricordo un Mastella ragazzo che a Benevento presentava Aldo Moro, che teneva nel teatro principale della città il suo ultimo discorso politico (poi ci fu il rapimento, cui seguì la tragedia che ben conosciamo), e ricordo il giovane democristiano che presentava, con emozione, Aldo Moro. Erano altri Erano altri tempi, in cui Moro si sarà interrogato tante volte se fosse utile o no andare in quello che era un territorio già allora abbastanza gelosamente custodito dai predecessori dell'onorevole Mastella nella gestione territoriale di quella Regione; Moro ci avrà pensato a lungo. Ricordo, come se fosse accaduto ieri, quel discorso, che fu molto più bello di quelli che ho letto poi negli atti successivi Moro tenne ai Gruppi parlamentari della Democrazia Cristiana, i discorsi con cui convinse la Democrazia Cristiana alla solidarietà nazionale; poi vennero i Governi del presidente Andreotti, in cui il presidente Prodi era Ministro dell'industria. Altri ricordi, altri scenari, il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, Mastella che spiegava nel *bunker* di Ceppaloni quello che stava avvenendo, la discesa in campo di Berlusconi, poi ancora l'UDR di Cossiga, il suo ripensamento, e la signora Sandra lì che faceva politica, mescolando valutazioni, che già allora erano ascoltate, con l'intrattenimento anche conviviale degli ospiti. Voi direte: che c'entra? C'entra: dico - guardando quei banchi che sono della vostra maggioranza - "ci azzecca", perché quei due non più ragazzi hanno creduto nei miei stessi valori, poi gli scranni parlamentari possono essersi ribaltati (nel caso di Mastella si ribaltano anche frequentemente), quindi tutto è provvisorio, mai come in questo momento, ma i valori da cui veniamo sono gli stessi, le storie personali che abbiamo vissuto sono le stesse. Il mio discorso, dunque, oggi non è di solidarietà, non so se pelosa o imberbe, ma di difesa di un'identità, di una storia e di uno stile. Sandra e Clemente Mastella sono due democratici cristiani, sono due persone per bene, guidano un partito che non rappresenta il mio modello - lo dico con sincerità - né di stile né di reclutamento del consenso, ma non è l'associazione a delinquere che vuole tratteggiare il mattinale di una procura di provincia. Rispetto a questo, signor Presidente del Consiglio, credo che la scelta tocchi a lei. Non, per carità, di promuovere le azioni che pure la Costituzione assegna, come

delle telefonate di raccomandazione. Ma guardate quanto è strano il corso e il ricorso storico che volge sempre, nella replica vichiana, la seconda edizione non più in tragedia ma in commedia. Oggi è la commedia della tragedia di Tangentopoli che, anche allora, cominciò con l'arresto di mezza Giunta regionale lombarda, guarda caso, inquisita e processata per aver fatto una riunione di spartizione dei *manager* delle ASL (col tempo, sono stati tutti assolti). Tanti anni dopo parliamo ancora di questo.

in uno qualsiasi dei tre ruoli che oggi ricopre. A lei tocca decidere se sopravvivere - e la vedo complicata, a giudicare dalla giornata - o rilanciare, che è ancora una facoltà, un diritto e una possibilità di questo Governo. Credo che vi sia oggi nel Paese il clima che Manzione negativamente ha denunciato e che invece io positivamente descrivo: il Popolo delle Libertà e il Partito Democratico sono due fatti politicamente nuovi. È innegabile che vi sia la possibilità di varare assieme una legge elettorale, forse una riforma costituzionale. Oggi dico al Neoministro: la famosa separazione delle carriere è un ripensamento della giustizia che sicuramente allontanerebbe il rischio di una replica di giornate come queste. Il mio è un discorso leggermente diverso dall'invocazione abbastanza consueta di tornare a casa anche perché conosco e frequento Bologna e dall'esterno conosco anche la sua casa, signor Presidente del Consiglio, quindi non credo sia una dannazione rispedirla lì: è una bella casa. Il tema di oggi è un altro: o noi facciamo le cose di cui il Paese ha bisogno (e possiamo farle assieme: Berlusconi, ancora pochi attimi fa, alla Camera, ha rilanciato questa disponibilità) o è inevitabile che il ricorso immediato alle urne sia l'unico rimedio. Questo Governo succede a tanti altri Governi, costituiti sul teorema della seconda Repubblica per cui bisognava fare qualsiasi cosa perché così Forza Italia e Berlusconi nel frattempo si scioglievano. Mi permetto di farvi notare per l'ultima volta che Forza Italia ha preso il posto del partito di cui rivendico la ragione sociale ormai da tre lustri. Ha davanti a sé ancora cinque anni (di Governo o di opposizione: ma ci sarà ancora per cinque anni), perché dubito che si scioglierà prima della prossima legislatura. In attesa, voi vi ammucchiate, vi riammucchiate, vi rilanciate, stentatamente vivacchiate in attesa che si sciolga un partito, un *leader*, una coalizione che invece sta tornando al Governo o comunque ha la massima popolarità sulle ali degli insuccessi di questa maggioranza e di questo Governo. Allora ribalto e replico a voi: attenti, perché io amo la politica e non vorrei che alla fine del percorso di questo Governo non trovassimo più la sinistra e, per questa valida classe dirigente che lei comunque, signor Presidente, ha con sé in tanti elementi al Governo, rimanesse solo la speranza di una telefonata a Bassanini per un reingaggio di Sarkozy.

è inutile negare che sono giorni molto complessi in cui tutto il Paese è sottoposto ad una grande pressione emotiva, in cui esiste anche il rischio di pesanti lacerazioni nel tessuto sociale del Paese. In questa complessità si è inserito un momento difficile per il ministro Mastella. E noi, come Gruppo Per le Autonomie, vogliamo esprimere solidarietà alla persona e al politico Clemente Mastella e solidarietà al partito dell'Udeur che è stato colpito da questa indagine giudiziaria. peraltro anche un apprezzamento vero e non formale per la decisione pressoché immediata del ministro Mastella di rassegnare le dimissioni, per affrontare serenamente il tema giudiziario che ha di fronte.

ciò auspicando che la situazione si chiarisca il prima possibile e che quindi anche il ministro Mastella possa ritornare alle sue funzioni, cosa che davvero ci auguriamo al fine di rasserenare il clima; il Paese ha bisogno di un clima più sereno e di maggiore coesione. Tuttavia, il fatto in sé e le modalità con cui l'azione giudiziaria si è dispiegata nelle ore della giornata di ieri non neghiamo abbiano suscitato molti interrogativi e, se vogliamo chiarezza, questa deve esserci davvero su tutto. Il tema ha riaperto anche la questione della democrazia, perché il rapporto fra potere politico e potere giudiziario è l'essenza vera della democrazia di un Paese, molto di più del rapporto fra potere politico e altri poteri dello Stato o tra potere politico e corpi sociali.

perché tutti i cittadini si sentono ugualmente garantiti e tutelati nei loro diritti sia con riferimento alla giustizia penale che civile. Sappiamo quanti danni anche economici arreca lo Stato con la sua lentezza e incertezza di giudizio,

che troppo spesso in questo Paese si sta perdendo ai diversi livelli, vada pienamente recuperato, ridando un ruolo alla politica, *in primis*, ridando fiducia ai cittadini, in modo che ci sia la possibilità di costruire davvero un tessuto sociale in questo Paese e si possa ricostruire un orizzonte di valori condivisi.

da lì dobbiamo ricominciare per ridurre la conflittualità del Paese, per ridare speranza alla gente, per ritrovare un comune orgoglio di essere italiani, in un mondo che cambia velocemente ma del cui mutamento vogliamo essere protagonisti. Nella lacerazione complessiva della società, nella frammentazione cui stiamo assistendo, in cui spesso è davvero facile che i poteri travalichino e si sovrappongano uno sull'altro, dobbiamo ritrovare un ordine. Questo processo passa attraverso la politica, attraverso il Parlamento, che è il fulcro delle decisioni, e quindi qui, da quest'Aula, dal Senato e dalla Camera. Deve ripartire tra le forze politiche, recuperando il senso della dignità del posto che occupiamo,

Signor Presidente, questo è un momento di grande delicatezza per la maggioranza e il Governo. La vicenda che ha colpito il senatore Mastella si è abbattuta su di noi come un ciclone. Noi, Presidente, apparteniamo a una cultura politica che dà fiducia alla magistratura, vuole che essa sia autonoma e indipendente, che il potere politico non possa né debba condizionarla e che essa non possa né debba condizionare la politica. Contemporaneamente, è per noi fondamentale che la presunzione di innocenza resti fino al momento del giudizio, senza che sia emessa alcuna condanna, di ordine né morale, né politico. Presidente Prodi, attorno a noi spira un vento pesante di antipolitica (saremmo pazzi ad ignorarlo) ed è una antipolitica che ha più di una ragione. Ieri e oggi, per fare un esempio, abbiamo assistito ad un rincorrersi di dichiarazioni di solidarietà a Mastella funzionali solo ad attaccare la magistratura. Questo in uno Stato di diritto non è consentito e suggerisco a Mastella per primo di guardarsene. Chi appartiene alle istituzioni deve rispettare ogni potere istituzionale, senza invadere campi altrui. Chi appartiene alle istituzioni non può creare uno scontro tra poteri che sarebbe micidiale per la democrazia del nostro Paese. Non spetta a noi decidere se c'è colpevolezza o innocenza. Né spetta a noi (cosa curiosa questa) stabilire se i reati sono leggeri o pesanti o addirittura se quei reati non esistono perché fanno parte della pratica politica. Se questo è, bene che i giudici rompano tale pratica, perché essa è devastante per la vita civile di un Paese. Quella non è la pratica della politica, ma di una certa politica, dalla quale ci sentiamo distanti anni luce. Oggi la politica dovrebbe saper tacere. Sarebbe molto grave assumere un atteggiamento di difesa corporativa e ripetere gli attacchi che nel passato sono stati fatti alla magistratura, inammissibili e volgari allora, inaccettabili oggi. Abbiamo assistito a tentativi di imbavagliarla, a leggi *ad hoc*: non faccio l'elenco, sarebbe troppo lungo. Troppo spesso la politica si è ridotta a tifoserie: l'antipolitica nasce anche da qui, da questi atteggiamenti, dall'arroganza, dalla presunzione di intoccabilità. Noi temiamo, e molto, l'antipolitica, perché può portare a derive assai pericolose. Ma essa non si batte con il decisionismo oppure con leggi elettorali a misura di singoli partiti e con riforme della Costituzione a ciò funzionali. Tutto ciò l'alimenta. La casta (terribile termine, ma ormai di uso quotidiano) è esattamente questo: far coincidere le scelte politiche con propri interessi di partito o di potere. Leggevo ieri una dichiarazione dell'onorevole Pecorella. Così descrive la magistratura: "Un potere inquinato da alcune fazioni politiche senza limiti né responsabilità che decide di uomini, di Governi e dell'intero Paese, come ha fatto nel 1994 con il presidente Berlusconi, e come sta tentando di fare con l'attuale maggioranza". Ma stiamo scherzando? Sono frasi inqualificabili. Nessuno può escludere (nessuno di noi lo fa) che ci siano singoli magistrati che abusano o hanno abusato del loro ruolo, ma voglio dire all'opposizione che quando si criminalizza un'intera categoria si pratica l'esatto contrario del garantismo. Non ci sfugge che utilizzando la vicenda Mastella si stiano Non ci sfugge che utilizzando la vicenda Mastella si stiano scatenando calcoli politici che riguardano gli equilibri generali del Paese e dello stesso centro-sinistra. Ieri, ma anche oggi, dichiarazioni mettevano assieme la vicenda del Papa all'università, i rifiuti della Campania e (così è stato detto) l'inciviltà giuridica dei magistrati e chiedevano come soluzione un Governo istituzionale che metta assieme centro-destra e centro-sinistra. Tentativi che sono apparsi evidenti durante la vicenda della legge elettorale, negli accordi di vertice tra i due maggiori partiti. Mi auguro che tentazioni o disegni del genere siano sconfitti. Noi siamo stati spesso critici con il suo Governo, presidente Prodi. Forse lo saremo anche in futuro. Lo saremo ogni volta che l'azione politica ci parrà non adeguata alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori, dei pensionati; ogni volta in cui vedremo pericolosamente appannata la laicità dello Stato, un bene prezioso perché tutti si sentano rappresentati e riconosciuti come cittadini a pieno titolo indipendentemente dalla loro fede, dal loro orientamento sessuale, dal colore della pelle, dall'identità di genere.

il suo Governo è quello che rappresenta le posizioni più avanzate. Abbiamo appena iniziato un percorso che, dopo l'opera di risanamento dei conti del Paese, vuole ridistribuire reddito e risorse, che individua nell'aumento dei salari e delle pensioni il modo per ridare giustizia ai lavoratori; salari che sono insufficienti, in alcuni casi miseri, non per opera dello spirito santo, ma per responsabilità primaria delle imprese. Penso alla tragedia della Thyssen ed ai comportamenti inqualificabili del vertice aziendale. Penso al contratto dei metalmeccanici, alle lotte di quei lavoratori che sono costretti a fare per ottenere ciò che è un loro diritto, rimettendoci una parte del loro già misero salario. Penso che, dal 1993, i contratti vengono rinnovati sulla base di un'inflazione programmata che nulla ha a che vedere con l'inflazione reale, con la conseguenza di una perdita costante e continua del potere d'acquisto. Noi lavoreremo, presidente Prodi, perché questo percorso non venga interrotto da calcoli di potere, da egoismo di partiti, da lotte intestine e dia i frutti che i cittadini aspettano. Concludo, Presidente, dicendo che è davvero grave l'uso che certi settori stanno facendo della vicenda che ha colpito il senatore Mastella. Vogliamo che la giustizia faccia il suo corso, che Mastella possa liberamente difendersi e ci auguriamo, e gli auguriamo sinceramente, che dimostri la sua estraneità; ma la giustizia sia libera di fare serenamente il suo lavoro. Da parte nostra ostacoleremo, cari colleghi, in ogni modo, con tenacia, certo, con le forze ridotte che abbiamo, anche con una rinnovata battaglia delle idee, ogni scontro tra potere legislativo e potere giudiziario, così utile ad una certa politica.

dei temi della giustizia il mio Gruppo parlamentare preferisce parlare nell'occasione alla quale il Presidente del Consiglio ha fatto riferimento, quando saranno conosciuti, attraverso lo svolgimento della relazione sulla situazione della giustizia, nella nuova funzione di Ministro *ad interim* assunto dal Presidente del Consiglio, gli orientamenti e gli intendimenti del Governo. Credo sia bene, infatti, parlare di questioni così delicate al di là della concitazione del momento. Voglio dire soltanto che mi è piaciuto di più il Mastella di oggi di quello di ieri, sia perché parlava da Ministro e ha confermato le sue dimissioni, e quindi da uomo e da parlamentare che si difende, sia perché ha espresso un giudizio di fiducia nella magistratura italiana come istituzione, che noi, come Gruppo della Sinistra Democratica, ribadiamo fino in fondo. fino in fondo. Meno brillante, invece, è stato il tifo da stadio che ha accolto l'intervento di ieri del ministro Mastella; a me piacerebbe che sugli abusi della giustizia e sugli arresti arbitrari, il Parlamento manifestasse solerzia, entusiasmo nell'intervenire ed indignazione quando si tratta di un cittadino comune e non di uno di noi. Ma dei problemi della giustizia, ripeto, discuteremo la settimana prossima, dovremo presentare anche risoluzioni parlamentari, come prevede la legge. Un problema però c'è: se c'è una sovrapposizione tra compiti della magistratura ed attività politica, dobbiamo domandarci se la politica fa tutta la sua parte per evitare che questo accada. Non mi pronuncerò sull'inchiesta giudiziaria, non l'ho mai fatto e tanto meno intendo farlo in questa occasione quando non moltissimo si conosce. Si sa però che l'ipotesi accusatoria - l'ha confermato il collega Mastella questa mattina - riguarda la lottizzazione di posti di medici primari in Campania. Non so se è reato, non spetta a me accertarlo, spetta ai magistrati. Mi domando: ma noi cosa facciamo per porre fine a questo scandalo? Primari lottizzati! Non sto parlando di *manager* delle ASL, ma di primari lottizzati. In Calabria si ammazza per questo, per il potere nel sistema sanitario. Ma il male non è soltanto nel Sud, è in tutta Italia. E allora? Si fa o non si fa questa legge per riformare il sistema sanitario e per sottrarre la nomina dei medici che devono curare le famiglie italiane, i nostri figli, i nostri concittadini alle decisioni politiche o, quando la magistratura dovesse in questa o in altra occasione intervenire, ci limiteremo a dire: così fan tutti, perché proprio con me? Non si deve fare più così perché è vero che lo fanno tutti con sempre maggiore impudenza, ma è anche vero che così non deve essere. La collega Turco ha parlato di una proposta del Governo

La maggioranza in Senato è fragile, ma sappiamo che abbiamo un problema di consenso nel Paese. Lei, presidente Prodi, ha detto, ad inizio anno, che la grande questione aperta è la questione del carovita, la questione del reddito delle famiglie. Ebbene, riprendiamo con determinazione questo tema. Ci si deve occupare di tutto il resto, tutte questioni importanti (la legge elettorale, lo strumento con cui i cittadini scelgono i loro rappresentanti e i loro governanti, è importante, non è solo un problema dei partiti e dei loro interessi, che pure c'è),

C'è un livello di diseguaglianza sociale in Italia che la pone, fra i 15 Stati della vecchia Unione, all'ultimo posto insieme a Grecia e Portogallo. Interveniamo su questo.

che erano stati fissati nell'accordo di luglio 1993, quando è decollato il metodo della concertazione che ha consentito di avviare l'azione di risanamento del debito pubblico (siamo ben contenti che gli ultimi dati sono stati positivi), ma del quale finora hanno pagato il prezzo soltanto troppe categorie di lavoratori per le quali non si è applicata la parte che impone il recupero del loro potere di acquisto. Il Gruppo Gruppo di Sinistra Democratica è accanto agli operai metalmeccanici che in queste ore e in questi giorni attendono che si decida il loro avvenire, il loro futuro; attendono con 1.000-1.100 euro al mese con cui devono mandare avanti, a volte, una famiglia con un solo reddito. Così come attendono i pubblici dirigenti, i pubblici impiegati, e qui la controparte è il Governo. Dobbiamo superare l'idea che il pubblico sia tutto negativo, che i pubblici impiegati siano tutti fannulloni. Stiamo parlando di coloro che svolgono funzioni fondamentali, insegnanti ai quali è affidata l'educazione dei nostri figli, delle forze dell'ordine alle quali è affidata la sicurezza dei cittadini, dei Vigili del fuoco, degli infermieri. Ma riteniamo davvero che si possono mortificare queste categorie di persone? Riteniamo giusto che un insegnante di liceo (adesso ci si pone il problema del livello di istruzione), un padre di famiglia, a 50 anni, abbia il livello di reddito Quindi interveniamo, agiamo su questo: possiamo farlo; solo il centro-sinistra può avviare una politica sociale di redistribuzione del reddito, di recupero del potere di acquisto di salari e di stipendi, di lotta contro la precarietà del lavoro, di misure per impedire che si ripetano gli infortuni sul lavoro. Ecco, allora, superiamo anche quest'altro passaggio difficile. Noi accettiamo la soluzione che il Governo indica, ma soprattutto noi crediamo che il centro-sinistra possa e debba rilanciare la sua azione a partire dai problemi che stanno a cuore agli italiani, che sono due, fondamentalmente: la moralità della vita pubblica e la questione sociale aperta in Italia.

Signor Presidente del Consiglio, lei ha fatto un discorso breve e conciso in cui ci ha detto alcune cose che sapevamo già, perché ci ha raccontato che cosa ha fatto e cosa ha detto Mastella. Lo sapevamo, grazie. L'unica novità che ha portato il suo discorso è l'aver confermato in maniera chiara e inequivocabile la solidarietà al ministro Mastella. Non abbiamo ben capito che tipo di solidarietà, perché se è umana tutti quanti noi l'abbiamo data e tra l'altro non c'è nessuno meglio di me che possa comprendere le ambasce del ministro Mastella, non soltanto di questi ultimi tempi, ma per tutto quello che riguarda il suo Dicastero. Ma ci sembra pure che lei sia andato oltre e abbia accordato anche solidarietà politica, visto che l'ha invitato a rimanere al suo posto.

Paese. Si può girare intorno al problema quanto si vuole, si può minimizzare, ma resta un dato fondamentale: ieri il ministro Mastella, in un'occasione solenne

Il ministro Mastella ha dichiarato: «Mi dimetto, perché ho paura». Credo che non si sia mai verificato, in tutto il mondo democratico, un episodio di questa natura: un Ministro, un Guardasigilli che afferma di dimettersi non perché ha problemi di natura politica con il proprio Governo, né perché ha cambiato idea sulle linee programmatiche del Governo e della maggioranza, ma perché ha paura. anche che c'è un'emergenza democratica. Ha detto - ohibò! - quello che abbiamo sempre detto anche noi, magari senza aver paura, consentitemelo.

che forma un pacchetto di mischia soltanto intento a decretare l'umiliazione umana, mediatica e politica di chi è contro di loro; e che questo pacchetto di mischia ha agito in passato contro alcuni e oggi agisce contro di lui. Parole pesantissime. Parole che un suo Ministro, un Ministro del suo Governo ha addirittura definito eversive. del Consiglio, lei ci deve chiarire, deve chiarire al Paese come stanno le cose. Deve chiarire se ha ragione il suo ex ministro Mastella, che lei, fra l'altro, ha auspicato torni Ministro,

quello che ha detto il ministro Mastella, visto che non soltanto ha respinto le dimissioni, ma ha dichiarato che tiene l'*interim*, perché auspica che il ministro Mastella torni al suo posto, una volta chiarita la questione giudiziaria. Tutti quanti noi auspichiamo che il ministro Mastella possa uscire pulito dalla sua questione giudiziaria, ma se ne uscirà pulito significherà comunque che quelle parole che ha dichiarato probabilmente erano vere. se erano vere, dobbiamo domandarci, dobbiamo domandare a lei che oggi è Ministro della giustizia nonché primo Ministro, quali azioni intende intraprendere, quali norme intende varare affinché non vi siano più questi pacchetti di mischia: non ci

e i Gip, infatti, hanno un potere gigantesco che nemmeno noi, nemmeno lei, nemmeno il Presidente del Senato ha, ma solo loro: quello di mettere in galera la gente e di rovinare la vita delle persone. Quindi noi dobbiamo agire in questa sede affinché non ci sia nemmeno un caso di questa natura. I pacchetti di mischia, in un Paese civile, non devono esistere. io credo, lasciatemelo dire, colleghi, magari sbagliando, magari facendo una montagna di errori, però in buona fede, che la politica che ho cercato di portare avanti, che la Casa delle libertà ha cercato di portare avanti attraverso i disegni di legge governativi che sono stati, di volta in volta, proposti e approvati dal Parlamento, a cominciare dall'ordinamento giudiziario, è stata improntata proprio a questo fine. Voi avete fatto esattamente il contrario, perché se oggi c'è qualcuno che può fare il pacchetto di mischia e scorrazzare liberamente nel Paese, come dice il ministro Mastella,

c'è di peggio: se il ministro Mastella avesse torto e avesse ragione il ministro Di Pietro, che difende sempre a spada tratta e in ogni caso la magistratura,

caso mai accaduto nella storia del Paese nemmeno ai tempi più bui di Tangentopoli. Significa che lei oggi sta al Governo ed esprime solidarietà ad un partito di associati per delinquere, perché questo sta scritto nel capo d'accusa della procura di Santa Maria Capua Vetere. Le pare che un Governo possa stare in piedi su questi presupposti, signor Presidente del Consiglio? Lei deve dircele queste cose, deve dirci se ha ragione Di Pietro o se ha ragione Mastella. Non può sfuggire a questo quesito che è fondamentale per il Paese perché lei ama dire agli italiani che il Paese sta andando avanti verso «le magnifiche sorti e progressive», che l'economia andrà sempre meglio.

che gli investitori stranieri non guardano quasi mai il colore di un Governo ma guardano se il Paese è stabile. Noi abbiamo un Paese che, sotto la sua guida,

dove domina un governatore che è fondamentale per il sostegno al Governo, la spazzatura politica o giudiziaria - dobbiamo scegliere - di questo caso la spazzatura culturale della Sapienza. Questa è l'Italia che noi stiamo vedendo in questi giorni. *(Applausi dal Gruppo LNP)*. Io vorrei capire, signor Presidente, che cosa intende fare per farci uscire da questa *impasse*.

perché chiunque si intenda di giustizia sa quanto è pesante tale impegno. Lei non potrà dividersi: pensiamo soltanto agli impegni di natura internazionale che il Ministro della giustizia oggi ha in Europa, pensiamo a tutte quelle questioni ineludibili che ci sono al Ministero della giustizia. Vedo schierati i suoi Sottosegretari, evidentemente dovrà lasciare a loro la gestione del Ministero, questo credo che dovrà farlo. Lei ha detto che andrà avanti per una giustizia sempre più giusta, sempre più rapida, sempre più efficiente. Ma scusi, dove vive?

che stiamo peggiorando. Dopo i leggeri miglioramenti sulla velocità e sul numero dei processi che la macchina della giustizia italiana è riuscita ad esitare, stiamo tornando indietro. Per forza, già prima avevamo magre risorse, voi le avete tagliate selvaggiamente a cominciare dal decreto Bersani. Non lo dico io, ma il presidente della

Oggi lei ha l'occasione per fare questo regalo agli italiani: secondo i sondaggi farebbe felice otto italiani su dieci togliendo il disturbo e tornando a casa.

onorevoli senatori, signor Presidente del Consiglio, ascoltando le sue dichiarazioni iniziali e poi il dibattito che ne è seguito mi tornava alla memoria un romanzo che ho letto nei miei anni giovanili. L'autore è George Orwell il romanzo si intitola "1984". In un certo senso lo si può leggere come un'introduzione all'arte della politica, non della politica democratica, ma della politica di uno Stato totalitario e immaginario del futuro in cui la prima arte del politico è quella del "bispensiero". Il bispensiero è la capacità di affermare con eguale determinazione, con eguale decisione, con eguale ingenuità due proposizioni perfettamente contrarie tra di loro. Visto che sono in vena di citazioni, mi veniva in mente un articolo di un grande studioso italiano, Enrico Berti, sul valore ontologico del principio di non contraddizione in Aristotele. Se ci guardiamo attorno, e guardiamo alla sua maggioranza, signor Presidente, vediamo che una parte di questa - non solo il ministro Di Pietro, anche la senatrice Palermo in modo più *soft* sembra coltivare l'idea, quanto all'Udeur, che si pensava fosse un partito e invece era un'associazione a delinquere. È una posizione che per la verità, sia onore al ministro Di Pietro, egli ha enunciato prima dell'azione dei magistrati. I cittadini italiani sono propensi a credere a questa versione dei fatti, se non altro

Sembrava un partito, invece era un'associazione a delinquere. Una parte della sua maggioranza la prende così, anche con un certo sollievo. C'è bisogno di un capro espiatorio per Napoli che affonda sotto l'immondizia e il capro espiatorio naturalmente è un vecchio democristiano. È qualcosa che aiuta a ricostruire un certo sentimento di identità. Apro una parentesi: possibile che non vi sia alcuna iniziativa della magistratura sulla gestione dei fondi comunitari nella Regione Campania per far fronte all'emergenza ambientale? Possibile che non vi sia alcuna iniziativa della magistratura o se c'è va molto a rilento e viene continuamente rimandata, per far luce sulle responsabilità di una gestione ambientale largamente lasciata nelle mani della camorra e condotta con sovrano disprezzo della legge e delle regole del buon Governo? Pare che i giudici non si occupino di questo, ma della signora Mastella, sì.

e che sia inutile chiudere gli occhi davanti a questo fatto. Ogni giorno, i giornali ci riportano i bollettini di guerra di questo scontro istituzionale e ritengono che il ministro Mastella stia pagando per il fatto di non aver compiaciuto a sufficienza

timidamente affermato che il Parlamento ha diritto di fare qualcosa che non corrisponde esattamente alla lettera a quanto precedentemente determinato dall'Associazione nazionale magistrati. Non so quale di queste due versioni sia vera. Anzi, circola una terza versione, che tutti avete

se siamo sicuri che le pressioni per imporre il proprio uomo in una ASL siano state fatte solo dalla signora Mastella. I miei amici campani ne dubitano

Se queste scelte vengono fatte dalla politica, è ovvio che siano anche dentro un sistema di contrattazione politica, anche se magari più civile di quello di cui abbiamo testimonianza in Campania.

la politica ha perso il suo prestigio per l'iniziativa della magistratura e la controffensiva della politica ha fatto perdere il suo prestigio anche alla magistratura. Senza fiducia nella politica e nella magistratura, il Paese affonda e, di fatto, sta affondando.

dice assolutamente nulla perché, per mantenere insieme la maggioranza, lei non può dire nulla; deve dare l'impressione di condividere quello che pensano gli uni e quello che pensano gli altri. non è possibile perché in questo modo forse si sopravvive, ma non si governa il Paese e non si indica un percorso per uscire dalla crisi. Questo è quello che invece noi le chiediamo, cioè avere il coraggio di assumere la responsabilità di indicare un percorso.

non abbiamo motivo di avere paura tutti noi cittadini? come privilegio del parlamentare, ma come tutela della sovranità del popolo italiano perché, quando un parlamentare, un *leader* di partito o un Ministro della giustizia è intimidito, non è più in grado di fare ciò che in coscienza ritiene essere il mandato affidatogli dagli elettori. Non possiamo troppo facilmente liquidare la questione dicendo: perché non ci occupiamo delle prepotenze della giustizia anche contro il comune cittadino? Certo, dobbiamo farlo e qualcuno di noi ogni ogni tanto lo fa. In questo caso c'è però qualcosa di più: è in questione la sovranità del popolo italiano. Il presidente Prodi vuole Mastella ministro della giustizia condividendo il giudizio politico durissimo che ha dato Mastella, oppure no? E qual è il progetto del Governo per porre fine a questo scontro istituzionale? Senatrice Palermi, quello che cambia è solo che ieri lo scontro istituzionale era contro una parte soltanto, mentre adesso morde anche nell'area della maggioranza. Ne abbiamo avuto delle prove con il caso Unipol e con qualche altra avvisaglia. Adesso è toccato a Mastella. Qual è il percorso che indica il Presidente del Consiglio? Noi saremmo lieti di ascoltarlo, ma lui tace.

in quanto, appunto, provvisoria e accompagnata dall'auspicio politico di un prossimo ritorno del ministro Clemente Mastella al suo incarico ministeriale.

Non è nostro compito emettere giudizi di merito e non è nostro compito - è anzi gravemente sbagliato - utilizzare questa circostanza per rilanciare un conflitto tra istituzioni, tra politica e giustizia, di cui certo questo Paese non ha bisogno. Noi, signor Presidente, la pensiamo come lei e teniamo fermi alcuni capisaldi di un'impostazione generale. L'indipendenza e l'autonomia della magistratura, così come la separazione netta e forte dei poteri tra di loro, sono cardini essenziali del nostro ordinamento costituzionale. Quindi, nella fattispecie, per il senatore Clemente Mastella (al quale abbiamo espresso già la nostra solidarietà personale e umana) vale, come per ogni imputato, la presunzione di innocenza. Allo stesso tempo, è da respingere - noi lo facciamo con forza - la campagna aggressiva che in questa circostanza è stata scatenata contro la magistratura per delegittimarne preventivamente l'operato e per riproporre il sospetto di un ennesimo intervento ad orologeria che sarebbe, secondo molti colleghi dell'opposizione, all'origine dell'inchiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere. In sostanza, noi teniamo fermi, anche in questo caso, i cardini di una vera cultura politica garantista, che ci consente di porci in una collocazione diversa sia dal garantismo, un po' peloso e spesso d'alto bordo, che caratterizza una parte del una parte del Parlamento, sia dal giustizialismo sommario così diffuso - ahimè - anche all'interno del popolo di sinistra. Credo che anche in questa circostanza sia giusto attenerci a questi criteri, ma anche ad un altro elemento che voglio citare proprio a proposito delle questioni che concernono la giustizia italiana e visto che il presidente Prodi dovrà farsi carico - io credo e spero per poche settimane - dei problemi che la riguardano. È vero che la giustizia italiana ha gravi problemi e che vi sono inefficienze ed ingiustizie di vario tipo, ma spero spero di non apparire attardata rispetto a categorie del passato: questi problemi riguardano quella natura di classe che continua a caratterizzare il nostro ordinamento e la concretezza del sistema stesso della giustizia.

disgraziate (quelli che a Roma vengono chiamati gli sfigati). È possibile che un medio professionista non lo abiti mai? Credo che questo tratto non possa essere dimenticato: non è vero che le nostre carceri sono

rilevante: che questa circostanza non costituisca un'ulteriore e improvvida occasione per la politica di compiere la propria, ennesima, autoassoluzione! Non è vero che la politica è innocente: non parlo, naturalmente, della bufera giudiziaria che si è abbattuta su Clemente Mastella, ma di quella crisi della politica che continua a pervadere nel profondo questo Paese,

affliggono fino in fondo la nostra società. Lo citava già il senatore Salvi, lo cito anch'io: i dati diffusi questa mattina dall'ISTAT ci dicono che metà della popolazione italiana vive un'esistenza difficile e che una parte cospicua della medesima non ce la fa ad arrivare alla fine del mese. Signor Presidente, non vorrei che le difficoltà di questa vicenda ed i problemi, molto profondi, che stanno avvolgendo la nostra agenda politica, contribuissero a far passare questa realtà in secondo piano. Essa resta, a nostro parere, al centro della situazione politica e dei problemi che riguardano il suo, il nostro Governo. È in atto un'operazione per la quale è stato usato un termine che a non molti piace, come verifica, perché ricorderebbe il passato; è più corretto, forse, parlare di un confronto, ma io dico qualcosa di più: un rilancio vero e pieno della capacità d'azione e d'intervento di questo Governo. Credo che non vi siano più e siano scomparsi dal nostro orizzonte tutti gli alibi che finora hanno impedito al nostro Governo di esercitare fino in fondo

Penso che questa operazione che compiamo debba portare ad un punto (mi permetto una brevissima autocitazione): quando si tenne qua il dibattito iniziale per la nascita del Governo Prodi, ebbi a dire che era essenziale darsi come orizzonte uno slancio riformatore, portando fino in fondo quel mutamento e quel cambiamento della società italiana che in qualche modo chiudevano con la stagione non solo dei Governi di centro-destra, ma del berlusconismo.

che è apparsa una litania: se lo appare, non lo voglio neppure citare). Mi interessa un'altra cosa: che oggi siamo nella necessità e nelle condizioni di rilanciare realmente l'azione di questo Governo al di là

che una parte ampia del popolo italiano (quelli che lavorano, che vivono del proprio lavoro), si aspetta da noi e si aspetta dalla politica. Se non ci sarà questo cambiamento, credo che non solo questo Governo, ma l'intera politica rischia di perdere senso, rischia di continuare a precipitare in una crisi di sfiducia, di lontananza e di separazione che determinerebbe e sta determinando nel suo fondo la vera emergenza democratica di questo Paese. È necessario un pieno protagonismo della politica vissuta e partecipata da parte di un nuovo blocco un nuovo blocco storico per il cambiamento e la trasformazione in questo Paese. Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, desidero ringraziarla per la tempestività con la quale è venuto a riferire in Aula, ma mi consenta di esprimere una totale insoddisfazione per come lei ha tentato di liquidare la vicenda Mastella. Infatti, la sua sbrigativa comunicazione sulle dimissioni del Ministro della giustizia,

corretta, stante la situazione della politica italiana - non solo però ha il sapore del disbrigo di una semplice pratica burocratica, ma suona come offesa, quasi scherno nei confronti del Senato e del Parlamento. Non si tratta soltanto, signor Presidente, di un Ministro che si dimette per l'intervento della magistratura: il problema è più serio, riguarda i rapporti tra le istituzioni dello Stato e riguarda un'istituzione, la magistratura, che si sente aggredita, e riguarda i membri del Parlamento che spesso ritengono, a torto o a ragione, di essere spiati e condizionati nello svolgimento del loro lavoro. Da un Presidente del Consiglio, oggi anche Ministro della giustizia, ci aspettavamo qualche riflessione in più, lei invece ha tenuto a banalizzare, anziché a fare qualche riflessione in più. Lei, Presidente del Consiglio, non può far finta che la vicenda Mastella possa essere considerata e relegata a mero episodio ovvero ad un piccolo e provvisorio incidente di percorso: la vicenda Mastella, che ha portato alle inevitabili dimissioni, non è grave solo in sé, è molto più grave perché s'innesta in un contesto sociale pesantissimo, in cui è costretto a vivere da diversi mesi il nostro Paese. Lei non può sorvolare sullo sfascio etico e morale che passa attraverso la drammatica emergenza dei rifiuti in Campania ed arriva fino all'Università «La Sapienza» dove, in modo vergognoso, è stato impedito al Santo Padre di parlare in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico. Come non può far finta di non vedere lo sfascio che interessa, in maniera serissima, gran parte delle famiglie italiane, che si dibattono in difficoltà insuperabili per sbarcare il lunario ed arrivare serenamente e dignitosamente alla fine del mese. Basta aver ascoltato quello che ha detto pochi attimi fa un senatore alla sua maggioranza, il senatore Salvi. Non può eludere che tale sfascio civile e morale passa attraverso l'instaurazione di un clima di cui il suo Governo è anche responsabile, che sembra essere mirato a togliere la libertà personale ai cittadini. I cittadini si sentono controllati, spiati, quando vanno al supermercato, al cinema, al ristorante, in banca; si è instaurato un clima di grande disagio. Lei, presidente Prodi, non può far finta di nulla davanti al crescente senso di insicurezza sempre più diffuso che, nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine, vivono i cittadini italiani. In passato, sia durante la cosiddetta prima Repubblica che nella seconda sarebbe bastato molto, ma molto meno perché il Governo ed il suo Presidente prendessero atto della situazione nel nome della responsabilità e dell'interesse generale, facendosi da parte. Le voglio riconoscere, signor Presidente, una bravura, certamente non a fin di bene, ma sicuramente incommensurabile: lei riesce a tenere in piedi una coalizione che fa acqua da tutte le parti. Lei riesce in un modo veramente incredibile - ed i cittadini si domandano come faccia a far questo - da quasi due anni a governare questo Paese in condizioni veramente di grande disagio.

di poter restare chiuso nel fortino di Palazzo Chigi, tirando a campare e presentandosi in Parlamento soltanto nelle occasioni, come quella di oggi, in cui la Costituzione gliene fa obbligo e pensa di poterlo fare non per dare conto del suo operato, ma per fornire comunicazioni che appaiono, come ho detto all'inizio, semplici pratiche burocratiche ma, in effetti, nascondono tutta la sua arroganza ed un piano che rischia di portare il Paese nella nebbia sempre più fitta. Mi riferisco in particolare ancora alla vicenda Mastella. Anche lei, infatti, presidente Prodi, pur riaffermando la solidarietà all'ex ministro della giustizia, nei fatti e nelle sue affermazioni lo ha sconfessato politicamente. Ieri, oltre alla solidarietà personale gli aveva garantito anche quella politica fino al punto di respingergli le dimissioni mentre oggi ha scelto un'altra strada. Lei avrebbe dovuto chiarire se condivideva interamente la relazione del ministro Mastella resa alla Camera dei deputati. Mi riferisco, in particolare, alle dichiarazioni del ministro, laddove confessa di aver paura e se condivide ad esempio - leggo testualmente del discorso del senatore Mastella: «Si è di fronte ad un'opera di demolizione eterodiretta, tesa a scardinare il presunto sistema di potere». Ma sotto un suo Governo siamo arrivati a questo punto? Condivide anche ciò che ha detto Mastella ieri: «In questa giornata è dato solo prendere atto di questa scientifica trappola che mi è stata tesa mediaticamente prima e giudiziariamente dopo in modo vile ed ignobile». Chi ha teso la trappola a Mastella e a tutta l'Udeur? Certo non potevano essere le forze di opposizione che non gestiscono né il Governo né il sottogoverno. dopo quasi due anni di suo Governo, la magistratura è quella dipinta dal senatore Mastella? Allora lui è stato a capo per due anni di un branco di delinquenti, così come definiti da Mastella ieri ? Tutto questo è accaduto in questi due anni! Anche noi a volte siamo stati critici perlomeno nei confronti di una parte della magistratura. Certamente non abbiamo mai partecipato alla criminalizzazione *in toto* di tutta la magistratura

A fianco di questa, certo, vi è una magistratura che preferisce i processi televisivi anziché lavorare nell'aula di un tribunale, ma non sapevamo che eravamo di fronte a una situazione come quella dipinta ieri dal suo Ministro, che ha rassegnato le dimissioni e che lei ha insistito tanto perché restasse al suo posto, e che ha detto: «Getto la spugna». Con il Governo Prodi ha paura persino il Ministro di grazia e giustizia! Ha ragione il collega Buttiglione: se ha paura il Ministro della giustizia, figuriamoci quanta paura hanno i cittadini italiani. Lei, signor Presidente, ha sorvolato, non ha chiarito nulla, e così facendo ha mollato Mastella ed ha riabbracciato, come spesso le è accaduto in questi quasi due anni, un altro Ministro che la pensa in maniera opposta a Mastella; mi riferisco al ministro Di Pietro. Ma è davvero possibile che l'Italia debba essere governata da un Presidente del Consiglio che sceglie i suoi alleati a seconda delle convenienze del momento? Lei ieri era con Mastella (e non parlo di "ieri" in senso generale ma

Non ci sembra che l'Italia possa ancora sopportare questa situazione intollerabile che assume i contorni del grottesco. Lei, presidente Prodi, se conoscesse ancora il significato della dignità e della responsabilità, dovrebbe uscire dall'Aula per recarsi al Quirinale. al Quirinale. Non credo che abbia avuto la bontà di ascoltare gli interventi di tutti i colleghi. Sicuramente non ha ascoltato

che questo Governo certamente non è amato nemmeno da coloro che lo votano. Infine, signor Presidente, lei ha detto che la prospettiva dell'*interim* limitata nel tempo, in attesa che il magistrato chiarisca velocemente. Non siamo al cinema, Presidente, non si occupa il posto con un soprabito in attesa che possa tornare il Ministro dimissionario. Lei è a capo di un'istituzione, l'istituzione più importante del Paese; non può pensare di ricoprire la carica *ad* *interim* e velocizzare la magistratura per far sì che il ministro Mastella possa tornare a svolgere

sulla definitiva situazione relativa alle dimissioni del ministro Mastella. Vorremmo ricordare e segnalare al Presidente del Consiglio come ormai noi si ritenga, come credo anche il Paese, questo Governo al suo epilogo.

Ormai non vi è giorno in cui questo Governo non dia al Paese una sua pena. Pensiamo alla vicenda dei rifiuti della Campania, che sta recando danni all'economia campana, ma anche all'immagine del nostro Paese, all'*export* di tutti i prodotti, nonché al turismo della Regione. alla politica estera. Non credo si possa ormai più rivendicare il primato della politica internazionale di un Paese guidato da un Governo che decide di trattare con i terroristi per la liberazione di ostaggi,

di una cultura cattolica che è stata sempre all'origine del primato della nostra coscienza e della nostra etica (mi riferisco al nostro Paese). Per quanto riguarda la vicenda Mastella,

Lei, ieri, dopo le denunzie, dopo l'intervento accorato, che molti italiani hanno seguito, del ministro Mastella, con cui egli lanciava delle denunzie significative (ancora più gravi in quanto provenivano dal Ministro della giustizia), con

lo ha fatto perché ci teneva ad evitare che si aprisse, come si è aperta, una crisi politica seria del suo Esecutivo, la cui stagione riteniamo ormai volga al termine.

al mondo della giustizia) che si faccia presto. Ebbene, non credo che ciò faccia onore ad un Presidente del Consiglio, che dovrebbe auspicarlo per tutti i cittadini e non solo per i suoi Ministri.

consentirà il ritorno in via Arenula di un uomo che ieri ha lanciato degli attacchi non indifferenti e gravi nei confronti di un certo funzionamento della magistratura. Diversamente, signor Presidente del Consiglio, dobbiamo darci delle risposte, dobbiamo essere conseguenti. La politica si lega, non si inventa, e lei non è uomo che inventi la politica, la conosce sicuramente molto bene. Questo dunque è il tema che le poniamo, questo è il tema che ci angoscia. Le parole del ministro Mastella ieri hanno colpito molti di noi. Non vogliamo entrare nel merito delle indagini giudiziarie: spetterà ai magistrati competenti. Tuttavia,

sia ormai oggettivamente reale perché colpisce esponenti di altre coalizioni, e quindi sia un fattore che comincia a diventare condiviso nella vita e nella politica del Paese, è un fatto che naturalmente ci fa riflettere attentamente e fa riflettere, mi lei. Vige però la sua strategia, quella della politica del giorno dopo giorno, pur di sopravvivere. Sappiamo che di qui a qualche mese lei sarà chiamato ad operare decine e decine di nomine di sottogoverno, per cui il suo interesse a sopravvivere, almeno fino a marzo-aprile, la farà da padrone. Vi sono nomine nell'ENI, nell'ENEL, alle Poste, alla Finmeccanica; in questo lei si è dimostrato bravissimo, nel gestire il potere istituzionale. Meno bravo, invece, nell'occuparsi di un Paese che è in declino: lo dicono gli osservatori internazionali, non lo diciamo noi. Nonostante l'aumento delle entrate fiscali, dovuto all'aumento della pressione fiscale al quale lo ha sottoposto, abbiamo un Paese che sta male: lo dicono i cittadini. È un Paese che soffre, un Paese che

ad assumere scelte impopolari pur di sopravvivere, pur di far durare il suo Governo. La sua è una politica economica che vede l'assenza di riforme strutturali di contenimento e di riduzione della spesa. Ormai questo Governo si avvita su se stesso; oggi (o ieri) la vicenda del ministro, o ex ministro, Mastella; mercoledì discuteremo qui la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Pecoraro Scanio, corresponsabile, assieme ai politici locali della Campania, della vicenda dell'emergenza rifiuti, di uno scempio sul territorio, consumato ad opera del suo Ministro, che in passato si è reso protagonista di quella politica del «no» a tutti i costi che ha arrecato grave danno all'economia del Paese e, paradossalmente, alla qualità della vita dei cittadini campani. Mercoledì torneremo a discutere di questo. Lo faremo con senso di responsabilità e siamo certi, caro signor Presidente del Consiglio, che anche mercoledì il suo Governo avrà le sue pene. Ci auguriamo, tuttavia, che quello sia l'ultimo giorno delle pene di questo suo Governo e che, con la sfiducia nei confronti del ministro Pecoraro Scanio, ella abbia ben compreso che occorre un sussulto anche di responsabilità: quello di invitare ella stesso i suoi Ministri a rimettere il mandato e, per lei, di recarsi al Quirinale, rimettere il suo mandato e tornare finalmente ad ad una nuova realtà, una realtà politica che ormai vogliono, auspicano, desiderano la stragrande maggioranza dei cittadini italiani, anche coloro i quali avevano votato per lei e oggi si sono pentiti di averlo fatto.

Prodi per l'attenzione, la tempestività e la correttezza istituzionale che ha dimostrato durante la vicenda che ha visto ieri le dimissioni del ministro Mastella, oggi confermate, e confermate insieme all'appoggio alla maggioranza che assiste il suo Governo. Vorrei fare alcune osservazioni di merito molto scarne; il dibattito è stato lungo ed i colleghi sono stanchi, ma non volevo lasciare trascorrere inutilmente questa occasione. Ho notato, ascoltando con attenzione il dibattito di oggi, ma in particolare gli interventi dei colleghi dell'opposizione, uno scarto molto forte rispetto a quello che è accaduto ieri nell'Aula della Camera e in quest'Aula. Ieri, nell'Aula della Camera, l'intervento del ministro Mastella, oggi così contestato, chirurgicamente sezionato, è stato oggetto di prolungati, prolungatissimi e vivacissimi applausi da parte dei colleghi del centro-destra. Ieri, in quest'Aula, ho sentito con le mie orecchie, e ciascuno di noi ha osservato, i colleghi dell'opposizione che con un gesto di generosità - devo dirlo - hanno dimostrato piena solidarietà al ministro Mastella. Oggi sono cambiati i toni: non mi stupisco, capisco anche che la giornata di ieri ha riaperto ferite ed in qualche modo, lo dicevamo nel ragionare comune, abbiamo agitato fantasmi. Primo fra tutti, quello di un conflitto tra la politica e la magistratura; dirò di più: ha riportato alla luce quella insofferenza, quella intolleranza nei confronti di un controllo avvertito molte volte come invasivo, come prepotente, come non arginabile. Intolleranza ed insofferenza che hanno segnato la storia politica italiana e negli anni scorsi hanno condotto a modifiche legislative che non abbiamo condiviso, alcune delle quali la Corte costituzionale ha dichiarato essere travolgenti il principio di uguaglianza ed essere contrarie al nostro ordinamento. Tuttavia, forse quello scarto segnala altresì (anche oggi voglio fare delle notazioni positive) una una nostra collettiva difficoltà di tornare a fare i conti con una questione che ha appassionato il dibattito politico ed istituzionale italiano, che lo ha segnato tante volte in male, poche volte con un miglioramento

riferito e avvertito il timore che risorga il tema del conflitto tra politica e magistratura. Ne abbiamo discusso e anch'io ho affrontato il tema. Molti oggi, anche il presidente Berlusconi, sia pure sulla base della ricostruzione giornalistica della conoscenza dei fatti che tutti abbiamo avuto (ancora parziale, ovviamente), hanno messo in evidenza come esistano due livelli: la responsabilità penale, che sta ai giudici sindacare - noi diciamo - nel pieno, autonomo, indipendente esercizio della giurisdizione

condivido tale distinzione e so quanto pesi ogni volta che, ad esempio, la magistratura abbia da indagare sui reati contro la pubblica amministrazione, sui reati dei pubblici amministratori i quali agiscono legittimamente esercitando la prerogativa della discrezionalità amministrativa, che andrebbe, come è ovvio, orientata al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione.

la necessità di chiarire cosa significa, cos'è ciò che appartiene alla politica, anche perché, a mio parere, se chiariamo questo punto, se cerchiamo insieme di chiarirlo, in esso sta anche la possibilità di ordinare nuovamente il rapporto tra politica e magistratura, ma assai più più la possibilità di parlare credibilmente ai cittadini, di creare una relazione ricostruita con il Paese, di frantumare quell'idea, tornata tante volte in quest'Aula, in questi giorni, che la politica e le istituzioni siano - per dirla con una termine che non mi piace - il luogo del dominio incontrastato di una casta. È questo il punto che voglio approfondire - ve lo dico così, con parole semplici e che per noi tutti deve valere, a prescindere da ciò che può casualmente originare un'indagine penale (quasi sempre l'indagine penale nasce da una casualità, da una intercettazione, da un pezzo di carta, da una notizia raccolta):

non l'assoluto senza regola e senza sindacato, ma la responsabilità politica. Ieri, per parte sua, il ministro Mastella lo ha applicato questo principio, dimettendosi. Ma è un'applicazione ancora troppo scarsa quella che riscontriamo in questo Paese; mi riferisco al Paese come sistema, anche come sistema politico. La politica esigerà con forza e con ragione l'ambito delle proprie prerogative anche di fronte alla magistratura solo se sarà pronta ed efficace nel sindacare le responsabilità politiche, se sarà forte nella relazione con l'opinione pubblica e se saprà assumere decisioni e responsabilità sgombrando, appunto, il campo dall'equivoco che se non c'è un giudice non c'è responsabilità. È un principio molto impegnativo e molto costoso, lo so. Lo dico a tutti noi, ovviamente; lo dico ai componenti del Governo, agli attuali Ministri, ai Sottosegretari e al Presidente del Consiglio, ai quali va la mia assoluta fiducia.

sta nella libertà per i cittadini di scegliere la rappresentanza, anche di scelta precedente tornando a scegliere. Un principio moderno su cui si fondano tutte le moderne democrazie rappresentative. Questa è una delle ragioni per le quali vogliamo una nuova legge elettorale, una legge elettorale in cui si ripristini il rapporto tra eletti ed elettori l'elettore possa chieder conto, agire responsabilità nei confronti del proprio eletto, che non è scelto dai partiti, ma dal proprio libero voto e consenso. Oggi pomeriggio ho visto rincorrersi sulle agenzie le notizie di una polemica scoppiata tra i Gruppi di opposizione per le assenze che questa mattina avrebbero (ancora una volta) garantito la maggioranza e l'avrebbero favorita. Verrebbe da dire, riandando a quanto diceva il presidente Schifani: anche l'opposizione si avvita su se stessa. Ma non voglio parlare di questo polemicamente. Al contrario, voglio dire che non c'è stata alcuna intesa e lo dico con grande chiarezza. Non so a chi giovi, visto che l'accusa è stata rimpallata da un Gruppo di opposizione all'altro. Non c'è stata alcuna intesa tra il Gruppo del Partito democratico e qualunque forza di opposizione. Ancora una volta voglio guardare in positivo. Ciò che è accaduto ci consente, una volta di più, di guardare in prospettiva alla possibilità di dare all'Italia una legge elettorale ampiamente condivisa. Io, francamente, questa occasione non la sprecherei, perché anche questo, in parte, è un modo per esercitare insieme responsabilità politiche.